Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico l'on. Stefano SAGLIA. Cordialmente. *F.to* Silvio Berlusconi».

Colleghi, un attimo di attenzione, per cortesia. Devo riferire dell'esito della Conferenza dei Capigruppo di questa mattina. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario corrente ed il nuovo calendario dei lavori fino al 14 maggio. Resta confermato che nel corso di questa settimana, a partire da oggi pomeriggio, sarà discusso il disegno di legge collegato in materia di internazionalizzazione imprese e energia. Per tale provvedimento, ferme restando le ore complessive originariamente assegnate, si è proceduta a una nuova ripartizione dei tempi attraverso cessioni tra i Gruppi. Sempre del corso della settimana corrente, potrà inoltre essere inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea il disegno di legge concernente l'ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità (approvato dalla Camera dei deputati). L'esame potrà avvenire in occasione di eventuali sospensioni della discussione del disegno di legge collegato o anche con eventuale prolungamento degli orari delle sedute. Gli emendamenti a tale provvedimento, per il cui voto finale è richiesta la presenza del numero legale, dovranno essere presentati entro le ore 19 di questa sera. Nella seduta pomeridiana di giovedì 7 maggio non potranno aver luogo le previste interrogazioni a risposta immediata al Ministro del lavoro per un improvviso impedimento del Ministro, impegnato in una missione all'estero. Saranno pertanto poste all'ordine del giorno interpellanze e interrogazioni. Il calendario della prossima settimana, che prevede seduta con votazioni anche nel pomeriggio di giovedì 14 maggio, reca l'eventuale seguito del disegno di legge collegato, nonché la discussione della mozione Sbarbati sulla promozione della cultura ove non esaminata nel corso della settimana corrente - e della mozione Bianchi sulla Carta europea dei diritti del malato. La discussione generale del decreto‑legge sul terremoto in Abruzzo, ove concluso dalla Commissione, avrà inizio non prima della giornata di giovedì 14 maggio. Nel corso della prossima settimana saranno inoltre esaminati disegni di ratifica di accordi internazionali definiti dalla Commissione. Sottolineo che la prossima settimana l'Aula sarà convocata nella mattina di martedì, alle ore 11. Quindi, avremo una seduta antimeridiana di martedì e lavoreremo sino al pomeriggio di giovedì.

Il provvedimento è stato trattato in Commissione attraverso moltissime riunioni, per il fatto che si è dovuto tener conto anche dei lavori di Aula e della conversione in legge di alcuni decreti altrettanto importanti e significativi.

È stato un lavoro impegnativo, che in qualche modo ha costretto i lavori della Commissione industria a svolgersi con qualche lentezza. All'interno della Commissione c'è stato un proficuo confronto con l'opposizione,

stati accolti integralmente, altri hanno subito riformulazioni che in qualche modo hanno trovato il consenso della stragrande maggioranza della Commissione medesima. È inutile negare però che su alcuni aspetti le divergenze c'erano e ci sono. Spero proprio che nel confronto costruttivo che avverrà in Aula in questi giorni si potranno dirimere alcune questioni

Le imprese italiane lo attendono non soltanto per quanto concerne i distretti. Ricordo che l'articolo 1 in parte è stato anche ripreso in altro provvedimento (il secondo decreto anticrisi) e aggiungo che alcune altre parti dell'originario provvedimento trasmesso dalla Camera, l'Atto hanno subito degli stralci nel milleproroghe o in altri provvedimenti, per cui in qualche modo il testo della Camera è stato notevolmente modificato.

Mi riferisco alla contraffazione, che sappiamo essere un male che colpisce moltissimo l'industria italiana, sia quella piccola che quella del *made in Italy*.

che sappiamo bene quanto interessi non solo il mondo delle imprese ma anche quello dei cittadini. Anche su questo, invito tutti a ragionare in termini di pragmatismo e a considerare che questo Paese deve fare le sue scelte: meglio una scelta a volte sbagliata che una non scelta e il rinvio di alcune decisioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, non è la prima volta che ci troviamo di fronte a una situazione simile. Abbiamo all'esame un atto che viene considerato collegato alla manovra finanziaria; tuttavia, esso appare in larga misura orientato a riscrivere la politica energetica del nostro Paese, per provare ad assecondare il ritorno al nucleare, e contiene altre norme che è difficile non considerare stravaganti rispetto al contenuto che Il contesto dell'insieme appare nettamente disomogeneo contiene argomenti eterocliti: l'internazionalizzazione delle imprese, il bollo virtuale, l'autotrasporto, la *class action*. Ci dovrebbe essere un contenuto omogeneo, che incide su ambiti normativi precisi, e invece abbiamo un insieme eterogeneo che, a nostro parere, appare nettamente in contrasto con il principio della semplificazione della legislazione.

Sono costretto a ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione era stato fissato al 15 gennaio scorso. Dopo l'apposizione di questo termine, sono state convocate più di trenta sedute della Commissione in cui il Governo e il relatore hanno presentato, in maniera continuativa, disomogenea e disorganica, proposte emendative talvolta di grande rilievo dal punto determinando, attraverso un'applicazione forzata del Regolamento, una terribile disparità di mezzi. Infatti, il Governo e il relatore hanno avuto la possibilità di continuare a produrre a getto continuo emendamenti, quando invece tale facoltà veniva impedita ai parlamentari. Secondo la legge n. 362 del 1988, che ha riformato la legge di contabilità, ossia la n. 468 del 1978, i disegni di legge cosiddetti collegati devono contenere interventi connessi alla realizzazione della manovra finanziaria. In particolare, si prevede che lo *status* procedimentale dei provvedimenti collegati deve essere precisato in maniera tale che questi devono essere indicati nella finanziaria, ossia devono essere segnalati prima, in anticipo,

Il risultato è che si configura una politica di settore tutt'altro che equilibrata sul piano finanziario e nell'ambito delle risorse spettanti alle decisioni di natura finanziaria.

il raggiungimento dei saldi di finanza pubblica e di evitare che, nel corso dell'anno, vengano adottate misure che comportino il peggioramento della decisione di bilancio. A tal riguardo, riteniamo assai criticabile l'azione del Governo in ordine alla legislazione di spesa adottata in seguito alla manovra estiva, in particolare attraverso il ricorso reiterato alla decretazione d'urgenza che, di per sé, rischia di compromettere gli obiettivi dei saldi. Il provvedimento, nel suo insieme, ha quindi una notevolissima ambiguità di fondo, che si materializza in un testo prolisso, confuso e anomalo anche quanto a coordinamento legislativo. In particolare, alcuni articoli costituiscono una sorta di delega in bianco e, soprattutto, priva di oggetto. L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Tutto il contrario di come si configura il provvedimento al nostro esame. Ciò è complicato ulteriormente dal fatto che questo collegato possiede anche la caratteristica di di provvedimento *omnibus*, come si accennava all'inizio, contenente cioè elementi privi di connessione reciproca. Questo modo di procedere determina l'impossibilità da parte del Parlamento di esaminare in modo consapevole il contenuto delle disposizioni di delega, cioè quei vincoli che, nell'ottica del modello derivante dall'articolo 76 della Costituzione, dovrebbero costituire i limiti all'esercizio della funziona legislativa da parte del Governo.

Sulla base di tali ragionamenti critici, proponiamo pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1195.

Colleghi, posso chiedere maggiore attenzione, per cortesia? C'è un'Aula molto disattenta.

*(PD)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei partire dalla relazione del collega Paravia che auspica un confronto costruttivo che spero si possa finalmente realizzare nel contempo, rivolgere gli auguri di buon lavoro all'onorevole Saglia che ha assunto la carica di sottosegretario allo sviluppo economico. Presentiamo la questione sospensiva perché la legge di cui discutiamo solleva non poche perplessità, sia nel merito che nel metodo, nel metodo, che non sono state superate dall'esame svolto in Commissione; esame che ha impegnato in maniera appassionata tutti i componenti della stessa Commissione, dal Presidente al relatore, agli altri membri di maggioranza e minoranza. è mancata la possibilità di risolvere questioni ancora aperte che noi proviamo a sintetizzare in questo dibattito nell'auspicio che si possa tornare ad approfondirle visto che il provvedimento è di rilevanza strategica per il Paese, soprattutto in un momento di difficoltà In questo provvedimento si introducono numerose deleghe. Noi stessi, con i nostri emendamenti, abbiamo proposto di delegare il Governo a definire norme in talune specifiche materie e tuttavia le deleghe definite nel provvedimento sono prive, in numerosi casi, di principi direttivi e di criteri chiari, univoci, tanto da poter mettere il Parlamento nella condizione di esprimere un parere articolato sui progetti di decreti legislativo. Non è condivisibile, a nostro parere, la scelta adottata dal Governo in relazione alla modifica di decreti legislativi vigenti e alla deroga di norme vigenti. In particolare, ci riferiamo alle norme che regolano la tutela del territorio e la salvaguardia ambientale e le norme che dispongono, di fatto, la non competenza, l'esautoramento delle Regioni e degli enti locali dai procedimenti di natura autorizzativa. L'articolo 14, ad esempio, prevede una delega per l'adozione di decreti legislativi che dovranno indicare la disciplina per la localizzazione nel territorio italiano degli impianti di produzione dell'energia e degli impianti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, che si configura come priva di un oggetto definito, nonché formulata secondo principi e criteri direttivi privi dei necessari requisiti di tassatività e determinatezza, così come richiesti dall'articolo 76 della Costituzione, soprattutto nella lettura fattane da una consolidata giurisprudenza della Consulta e da ultimo, in particolare, dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 340 del 2007. La procedura indicata nel provvedimento per l'adozione dei futuri decreti legislativi sottrae alla competenza parlamentare il confronto con l'Esecutivo che, al contrario, dovrebbe essere ampio e approfondito, trattandosi di scelte di rilievo che modificano completamente lo scenario delle politiche energetiche del Altrettanto discutibile appare la scelta di affidare ad una delibera del CIPE la definizione delle tipologie di impianto per la produzione di energia elettrica da realizzare sul territorio nazionale, senza coinvolgere in tale procedura, sulla scorta di valutazioni della comunità scientifica e dei saperi tecnologici, le Regioni e gli enti locali e senza un parere vincolante del Parlamento. Il complesso delle disposizioni previste per il controllo della sicurezza nucleare e la radioprotezione delle centrali nucleari appaiono inadeguate a garantire la tutela dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente; la previsione dell'istituzione di un'Agenzia per la sicurezza non si rivela uno strumento adeguato a tale scopo. All'organo di vigilanza previsto per il controllo della sicurezza nucleare e la radioprotezione delle centrali nucleari non è assicurata la necessaria autonomia e i meccanismi di nomina espongono i membri ad ogni possibile forma di influenza da parte dell'Esecutivo e non garantisce l'autorevolezza e l'alta competenza necessaria. Per quanto riguarda il complesso delle misure per il potenziamento della rete infrastrutturale energetica, vengono proposte pericolose deroghe alla normativa urbanistica ed ambientale nonché semplificazioni alle procedure di autorizzazione, che esautorano di fatto le competenze attribuite alle autorità locali in materia di controllo e pianificazione del territorio esponendo le relative procedure alla incertezza derivante dalle opposizioni che scaturiscono dal mancato coinvolgimento delle comunità locali e dai ricorsi che inevitabilmente potranno essere proposti alla Corte di giustizia europea. L'ampliamento del *mix* delle fonti energetiche affidato alla ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma ed in mare evidenzia problematiche ambientali che non sono affatto trascurabili e che ignorano i princìpi elementari di precauzione, posti a tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente, criteri e procedure adottati in sede comunitaria. Forti preoccupazioni destano, infatti, sia le procedure per lo smaltimento dei residui delle prospezioni, sia i fenomeni di subsidenza che si possono verificare nelle aree marine e costiere, in particolare nell'area dell'Adriatico, fino ad interessare città storiche come Venezia e aree naturali come il Delta del Po. Destano altresì diverse perplessità l'introduzione di argomenti non attinenti al contenuto proprio del provvedimento; non si può in alcun modo condividere infatti la scelta di operare una rilevante riforma dell'azione collettiva risarcitoria, rispetto alla quale non sono mancate espressioni di rammarico, in particolare da parte dei cittadini rimasti vittime di frodi e delle loro associazioni, quindi dal condividere l'impostazione scelta dal Governo. In particolare, appare evidente l'irragionevolezza di una norma, come quella che limita l'esperibilità dell'azione collettiva risarcitoria ai soli illeciti verificatisi dopo il 30 giugno 2008. Altrettanto non condivisibile appare l'inserimento nel provvedimento di norme relative allo svolgimento del servizio ferroviario passeggeri in ambito nazionale, in materia di servizio universale, nonché di trasporto pubblico locale, che di fatto rinunciano ad acquisire l'autorevole orientamento del Parlamento esplicitato attraverso le Commissioni parlamentari competenti di merito e quindi rinunciano a quell'adeguato approfondimento che una materia tanto complessa e specifica avrebbe richiesto. Altro punto di forte criticità è costituito dall'articolo 24, che devolve al tribunale amministrativo regionale del Lazio la giurisdizione su tutte le controversie attinenti alle infrastrutture, agli impianti ed alle attività del settore energetico, dilatando irragionevolmente per l'intero territorio nazionale la competenza del giudice amministrativo, anche qualora siano denunciate lesioni dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. Sul punto la Corte costituzionale, nella recente pronuncia n. 191 del 2006, aveva chiarito che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si può giustificare solo in relazione ai principi costituzionali degli articoli 24 e 111, che mirano a concentrare dinanzi ad un unico giudice la tutela del cittadino rispetto alle modalità di esercizio della funzione pubblica. Tali norme, che derogano ai princìpi cardine del nostro ordinamento, non sono accettabili tanto più in quanto del tutto inidonee a perseguire il fine di garantire maggiore efficacia all'azione di contrasto alle attività connesse al corretto sviluppo del settore energetico, determinando soltanto un ulteriore ostacolo al lavoro della magistratura. Destano infine forti perplessità le disposizioni relative alla rimodulazione, al reindirizzamento ed al temporaneo blocco degli interventi per le aree sottoutilizzate e, in particolare, la rimodulazione degli interventi relativi ai patti territoriali, alla contrattazione negoziata e quindi agli accordi di programma, nonché per interventi di agevolazione a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Nel complesso, siamo di fronte ad una profonda revisione degli strumenti di incentivazione e di sostegno alle imprese che arrivano ad incidere anche sulle risorse, soprattutto quelle del e sulle competenze regionali in materia, tra l'altro affrontando tale operazione, da un lato, con una generica delega e, dall'altro, con un non coordinato meccanismo di norme di immediata applicazione. Per tutte queste ragioni, chiediamo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1195 sino alla data di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico- finanziaria per il 2010.

Il primo elemento da mettere in risalto è che, per l'esperienza di questi mesi di lavoro in 10a Commissione,

Il numero di emendamenti presentati dall'opposizione e in parte anche dalla maggioranza ha portato ad un approfondimento significativo di quasi tutte le parti costituenti il disegno di legge

è stato continuo in questi mesi e il numero degli emendamenti presentati rappresenta di per sé l'elemento fondamentale dello sforzo che è stato compiuto per approfondire diversi argomenti.

riporta come le deleghe sono relative a percorsi che comportano l'interazione sia con le amministrazioni locali sia, a volte, con lo stesso Parlamento.

un ponte verso l'innovazione e, contemporaneamente, verso l'utilizzo delle sorgenti di energia più avanzate, non dimenticando di introdurre elementi fondamentali per l'incentivazione delle sorgenti

una potenziale acquisizione dell'energia su un mercato molto più ampio, in particolare introducendo di nuovo in Italia l'importante percorso dell'energia nucleare.

nel disegno di legge per fare in modo che lo sviluppo italiano si basi su questo perno fondamentale: da una parte lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese e dall'altro l'acquisizione di nuove potenzialità in termini di sorgenti di energia e utilizzo

i quali abbiano meritato un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Questa regola esiste per una ragione molto evidente, che riguarda la sostanza della gestione della finanza pubblica e della politica economica di un Governo. Il disegno di legge viene dichiarato collegato perché il Governo e la maggioranza lo considerano essenziale al fine della realizzazione della loro politica economica e della gestione della finanza pubblica. Questa norma regolamentare copre e tutela il diritto del Governo e della maggioranza di poter realizzare la propria politica economica nel contesto finanziario fissato dalla legge finanziaria e dalla legge di bilancio. Ecco perché questa che alcuni colleghi considerano una stranezza, e cioè il parere contrario della Commissione bilancio su alcune parti di disegni di legge collegati, e naturalmente su alcuni emendamenti presentati a questo disegno di legge, è una norma regolamentare perfettamente coerente con l'esigenza di tutelare il diritto-dovere del Governo e della maggioranza di collocare le loro scelte di politica economica, fatte attraverso provvedimenti collegati, in un contesto finanziario certo e non modificabile da parte del Parlamento. Naturalmente, signor Presidente, questo implica che nemmeno emendamenti al disegno di legge possano essere votati, cioè dichiarati ammissibili, in Commissione e in Aula,

ci sono articoli, commi, anche molto rilevanti, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non tutti derivano dall'approvazione di emendamenti, come tali patentemente inammissibili se hanno avuto il parere contrario dalla Commissione bilancio, sia in Commissione sia in Aula, ma alcuni di questi articoli e di questi commi facevano parte del disegno di legge originario, nel testo riveniente dalla Camera, su cui immediatamente la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 Questo implicava non la possibilità, ma l'obbligo di realizzare un'operazione di ripulitura del testo da quei commi e da quegli articoli che non sono ammissibili perché scoperti finanziariamente. Signor Presidente, noi, a mio avviso, non possiamo procedere all'esame di un disegno di legge di cui fanno parte articoli e commi che erano - e sono tuttora -patentemente inammissibili in un collegato. Per questo motivo, non ho voluto porre la questione nella fase dell'iniziativa politica per la sospensiva, ma la pongo adesso sotto il profilo meramente procedurale. A mio avviso, si dovrebbe preliminarmente procedere sul testo uscito dalla Commissione attraverso operazioni di sua iniziativa, signor Presidente; non so quali, con precisione, ma potrebbe trattarsi di una sorta di dichiarazione come quella che si fa

Mentre ho memoria di iniziative rivolte a dichiarare collegato alla finanziaria, successivamente all'inizio dell'*iter*, un disegno di legge che originariamente non lo era, non ho memoria di un'iniziativa volta a dichiarare non più collegato un disegno di legge che, in origine, era nato come disegno di legge collegato. Il risultato, a mio avviso, è che ci vuole un'iniziativa della Presidenza

che l'Aula non può prendere in esame un disegno di legge licenziato dalla Commissione con al suo interno un testo che in parte, e per parti significative, era patentemente inammissibile in origine, lo è rimasto durante tutti i lavori della Commissione e lo è anche adesso. *(Applausi dal Grazie, La Presidenza ritiene che in questa fase sia opportuno quanto meno proseguire nella discussione generale e concluderla, possibilmente, entro questa sera o domani mattina.

necessaria e indispensabile una sospensione della discussione di questo provvedimento per consentire alla 5a Commissione di concludere il proprio lavoro sia sugli emendamenti che sul testo. È un atto dovuto. Le assicuro, senatore Morando, che a conclusione del lavoro della 5a Commissione, e quindi dei pareri resi sia sul testo che sugli emendamenti, questa Presidenza adotterà

abbiamo deciso che in presenza di sospensioni d'Aula dovute alle esigenze dei lavori della 5a Commissione si sarebbe esitata un'altra leggina - quella che consente il diritto di voto ai malati e agli inabili

disegno di legge n. 1195 finiremo in un tempo molto breve. La questione posta dal senatore Morando ha delle altre implicazioni, ma sul testo finiamo in tempi brevissimi.

per quanto riguarda lo specifico del testo degli emendamenti, la decisione che lei sta prendendo va benissimo. Io, però, vorrei insistere su un punto che a me sta molto a cuore, perché non vorrei che si stabilisse un precedente che per la decisione di bilancio del Senato risulterebbe esiziale, cioè che sia possibile proceduralmente, mentre si discute di un disegno di legge collegato, mettere in votazione

È come se durante la legge finanziaria lei, Presidente, e il Presidente della Commissione bilancio non poteste dichiarare inammissibili gli emendamenti scoperti. Vorrei che fosse colto il punto. Sul disegno di legge in questione vediamo come fare, ma c'è un problema più di fondo: un testo che contiene delle parti che in nessun modo avrebbero dovuto arrivare all'esame dell'Aula, e nemmeno alla votazione della Commissione, perché sono inammissibili, non perché lo dico io, ma perché lo dice il Regolamento del Senato.

se non attraverso una procedura che violi il principio che ciò che è scoperto nel collegato è inammissibile. E questo - insisto - non perché è il mio parere, ma perché è quello che inoppugnabilmente è scritto nel Regolamento del Senato.

un qualche problema di rapporti, ma non può accadere una seconda, perché è chiaro che costituirebbe un precedente lesivo del diritto non dell'opposizione, ma del Governo e della maggioranza a tutelare in Parlamento i loro disegni di legge collegati da iniziative di sfondamento degli equilibri di bilancio. È una questione assolutamente fondamentale per la politica economica e per la gestione della finanza pubblica. *(Applausi della

la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

lavoro incessante e paziente svolto dalla Commissione che lo ha esaminato per competenza e per merito, disegna un serio, organico e coraggioso intervento di politica economica.

non solo per le riflessioni sull'importanza e sulle ricadute dei singoli dispositivi svolte dal relatore, che ha avuto l'arduo compito di riassumere sinteticamente...

un provvedimento mediante il quale il Governo formula in maniera chiara, benché articolata, la filosofia e le priorità che esso persegue in materia di politiche per uno sviluppo possibile, sostenibile, ed io aggiungerei altri due aggettivi, che considero importanti: prossimo, cioè vicino, e responsabile, che è quanto mai importante in questa fase. È l'assunzione di responsabilità che il Governo di Silvio Berlusconi, responsabile di come affrontare la crisi e di come traghettare il Paese oltre la crisi. quello all'esame dell'Aula è un testo migliorato dalla Camera e ulteriormente potenziato dalla Commissione di merito in questo ramo del Parlamento, che esprime la logica con la quale il Governo intende intervenire sulla struttura economica e produttiva del Paese. E non è un caso la presenza del ministro Scajola in Aula, che segna l'attenzione e la puntualità di questo Governo verso uno dei settori vitali del nostro sistema Paese. Una logica qualitativa - l'opposizione potrebbe dire velleitaria, ma oramai siamo abituati a questo *leit-Motiv*, altro che sospensive, altro che pregiudiziali! - espressa da questo espressa da questo Governo in tutte le misure messe in campo, che ricomprende diversi ambiti di intervento, tutti esiziali, tutti fondamentali: la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione, la proprietà industriale, l'energia, le società cooperative e - tema che sta a cuore a tanti di noi - i consumatori, il ruolo e la difesa dei cittadini e dei consumatori. Una logica qualitativa ispirata a concetti e princìpi molto chiari: razionalizzazione e semplificazione di settori e normative. Penso agli interventi sul sistema degli incentivi e alle agevolazioni per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, ovvero agli adempimenti procedurali e alle certificazioni per le imprese; intervento qualificante su strutture peculiari del nostro sistema produttivo. Penso inoltre alle disposizioni per la configurazione e la razionalizzazione dei distretti e delle reti di imprese;

pensando alle numerose norme che riguardano il settore dell'energia. E ancora, la valorizzazione delle nostre produzioni più tipiche; penso alle innovazioni in materia di tutela penale, dei diritti di proprietà industriale ovvero a quelle sul diritto d'autore o a quelle anticontraffazione. Tutte misure finalizzate a salvaguardare, a sostenere e a migliorare le condizioni entro le quali lavora il cosiddetto *made in Italy*. all'apertura e alla trasparenza dei mercati e alla tutela dei diritti dei cittadini. Credo che per la prima volta vi sia un intervento per l'adozione di una legge annuale esplicitamente riferita al mercato e alla concorrenza, e io ringrazio il ministro Scajola per questo, ci dà la misura della modernità di questo strumento, di questo impianto normativo, ampio, difficile, non sempre di facile lettura, che però mostra e dispiega tutta la sua forza. Così come non possono sottacersi gli interventi previsti in materia di liberalizzazioni di alcuni settori (quelle vere, non quelle fittizie) o quelle per il riordino di competenze di alcune *Authorithy* o, ancora, quelle, apparentemente più semplici (spero che qualcuno di noi non voglia definirle populistiche), sulla riduzione e la conoscibilità del prezzo dei carburanti o, infine, alla *class action*. Una logica qualitativa ispirata anche alla risolutezza. Ritengo, infatti, che questo sia un provvedimento coraggioso (come affermato dal sottosegretario Urso alla Camera), perché affronta, fuori da schemi ideologici e fariseismi (uno dei mali del nostro sistema politico), uno dei nodi cruciali del nostro sistema: la dipendenza energetica. C'è per la prima volta il riferimento esplicito all'energia nucleare alla possibilità di considerarla uno strumento a disposizione del Paese nel suo complesso. È il vecchio sogno di Enrico Mattei, ministro Scajola: autosufficienza perseguita con realismo e coraggio, l'orgoglio di essere un Paese tra i grandi, un modello da esportare e non una colonia. Un Paese che ha saputo produrre, anche in questi momenti difficili, esempi come quello della FIAT, dei distretti, che ci è copiato da tanti Paesi, delle piccole e medie imprese, del Nord‑Est, dell'aumento delle partite IVA. In un momento così tribolato, ha fatto bene il ministro Tremonti a mettere in evidenza come, in questo Paese, qualcuno ha ancora la voglia ogni mattina di lavorare, di inventarsi un'impresa. E 170.000 nuove partite IVA sono il segno di una grande vitalità, di un Paese che non si arrende, che non smette di sperare nella sua grande radice culturale, quella dell'impresa, spesso legata alla famiglia, di sicuro legata al suo territorio. Con questo provvedimento il il Governo intende fornire risposte ad alcune questioni che riguardano gli aspetti strutturali del nostro sistema economico e produttivo, cioè quelli reali della nostra economia. Vorrei ricordare che il disegno di legge in esame è un provvedimento collegato (lo diceva bene prima il senatore Morando, che ci ha richiamato anche ad alcune questioni formali e sostanziali),

per affrontare questa crisi. Prima ancora - ripeto - che essa dispiegasse i suoi effetti. E mi sembra in corso di completamento un'intera manovra, che comprende anche quel federalismo fiscale che abbiamo approvato solo qualche giorno fa. In tal senso, mi sembra che questo disegno di legge possa confermare *ex* *post* una caratteristica che si era posta evidente *ex ante*, cioè uno strumento che può considerarsi il *pendant*, il necessario completamento degli interventi adottati, anche più recentemente, per contrastare la pesante crisi finanziaria internazionale. Spero che le valutazioni - che legittimamente possono differire - dall'altra parte di quest'Aula siano lontane dalla strumentalità e da critiche cosiddette a prescindere.

quanto conosce il sistema economico italiano reale e quanto è capace di fare per migliorarlo, per adeguarlo, per sostenerlo, abbattendo il *moloch* della burocrazia inutile, che tanto pesa sulle spalle del sistema Paese, delle sue imprese, dei suoi lavoratori e dei suoi cittadini.

(auguri al sottosegretario onorevole Saglia, che vediamo qui per la prima volta), colleghe e colleghi, sul complesso del disegno di legge Senato n. 1195 al nostro esame, composto di ben 33 articoli, mi limiterò nel mio intervento a considerare unicamente tre articoli: gli articoli 14, 15 e 17, che nel loro insieme individuano le disposizioni necessarie per la reintroduzione nel nostro Paese dell'energia nucleare. Un grande fatto. Lasciatemi dire che tale reintroduzione suscita in me una profonda soddisfazione. Sono ingegnere nucleare e ho avuto il privilegio di esercitare davvero questa professione non l'hanno fatto molti in Italia - per oltre ventisette anni, maturando in tale esercizio la certezza della validità di questa tecnologia e, in particolare, della sua assoluta sicurezza. Ma insieme a questa soddisfazione permane in me il rammarico per il gravissimo errore compiuto dalla nostra dirigenza politica alla fine degli anni Ottanta, quando, successivamente all'esito del *referendum* del novembre 1987, venne deciso l'abbandono della tecnologia elettronucleare. E ciò nonostante gli importanti investimenti già fatti (ne ricordo solo uno, quello relativo alla centrale elettronucleare di Caorso, 850 megawatt elettrici, già perfettamente funzionante all'epoca); nonostante l'evidente necessità per il nostro Paese, dipendente dall'estero per oltre l'85 per cento del proprio fabbisogno energetico, della massima diversificazione energetica; nonostante il fiducioso ricorso all'energia nucleare effettuato da tutti gli altri principali Paesi d'Europa, Francia in testa, e poi Germania, Spagna, Gran Bretagna. Ancora oggi la percentuale di energia elettrica ottenuta per via nucleare nei 27 Paesi dell'Unione europea - tra cui l'Italia che non produce energia elettronucleare - ammonta al 30 Purtroppo i giornalisti e i guru della comunicazione esperti nella denuncia di sprechi e cattive gestioni nell'ambito pubblico (denuncia encomiabile, sia ben chiaro) non si sono minimamente dedicati alla valutazione e men che meno alla pubblicazione delle nefaste conseguenze di quella decisione e dell'enorme danno che ne è derivato (e continua a derivarne) ai nostri cittadini e alla nostra economia. Al contrario: vi è stata per venti lunghi anni una martellante intossicazione mediatica, ideologicamente ispirata, tesa a misconoscere ogni pregio dell'energia nucleare, anzi a demonizzarla, onde impedirne per sempre una sua reintroduzione. Ancora oggi non si contano i Comuni che esibiscono al loro ingresso l'insegna «Comune denuclearizzato» (come, ad esempio, il Comune di Arcore). Tale perniciosa azione di disinformazione continua purtroppo anche ora. Ne è esempio la trasmissione "Report" di domenica 29 marzo scorso su RAI 3, in prima serata, dedicata appunto al nucleare.

(in base all'articolo 21 della Costituzione i cittadini hanno diritto di ricevere un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata), in questa trasmissione si sono sistematicamente interpellate persone non aventi specifica competenza nel settore nucleare e ignorate le istituzioni nazionali e internazionali competenti nelle materie trattate; si sono qualificati come indipendenti soggetti e organizzazioni oggettivamente orientati in senso antinucleare; si sono veicolate affermazioni destituite di fondamento scientifico; il tutto senza il minimo contraddittorio. Passiamo adesso all'esame del testo di legge alla nostra attenzione. L'articolo centrale per la reintroduzione della produzione elettronucleare nel nostro Paese è l'articolo 14. Tale articolo delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più (saranno certamente più d'uno) decreti legislativi riguardanti le principali problematiche relative a tale reintroduzione. Di grande importanza è la coraggiosa previsione di un'autorizzazione unica (a seguito di procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate) per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettronucleare, previsione che toglie una cospicua incertezza sui tempi di effettiva entrata in funzione di tali impianti nucleari, contribuendo in modo rilevante a ridurne i costi. Di grande importanza è anche la previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni da autorità di sicurezza competenti di Paesi membri dell'OCSE o di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali siano considerate valide in Italia. Ciò consentirà alla nostra Agenzia per la sicurezza nucleare di avvalersi delle approfondite analisi di sicurezza svolte da Agenzie di sicurezza di altri Paesi, aventi ben maggiore esperienza, senza doverle rifare. Di grande rilevanza sono anche le disposizioni riguardanti la delicatissima scelta dei siti nucleari (sia i siti su cui installare le centrali nucleari, sia i siti da adibire a stoccaggio temporaneo o deposito definitivo dei rifiuti radioattivi). Al riguardo, i decreti legislativi prevederanno la possibilità di dichiarare i siti «aree di interesse strategico nazionale»; definiranno i requisiti tecnici dei siti necessari per soddisfare le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente; definiranno le misure compensative alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito; determineranno le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle intese con i diversi enti locali coinvolti. L'articolo 14 prevede inoltre che saranno individuati, sempre per decreto legislativo, gli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica. Si tratta di un'importante disposizione a favore del produttore di energia elettronucleare, perché consente la riduzione a costo certo e limitato di un costo incerto che potrebbe essere anche assai rilevante. Nei decreti legislativi di cui all'articolo 14 saranno altresì previste le modalità attraverso cui i produttori di energia elettronucleare contribuiranno ad un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e per il trattamento e smaltimento finale di rifiuti radioattivi al termine della vita operativa degli impianti.

volta ad evidenziare in particolare sicurezza ed economicità di tale forma di energia, sia opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni direttamente coinvolte. Tali campagne informative sono, a mio avviso, particolarmente opportune, data la sopra richiamata profonda intossicazione mediatica antinucleare a cui la popolazione italiana è stata sottoposta per oltre vent'anni. I decreti prevederanno anche le modalità del finanziamento di tale azione informativa. Di grande importanza, sempre relativamente all'articolo 14, il comma 3, volto a limitare l'incidenza dei provvedimenti giurisdizionali davanti agli organi di giustizia amministrativa riguardanti la realizzazione delle opere concernenti il settore dell'energia. Si estendono così, per sostenere la fiducia degli operatori economici, anche al settore dell'energia modelli processuali già sperimentati dal legislatore in altri settori e ritenuti legittimi dalla Corte costituzionale. L'articolo 15, comma 1, riguarda le modalità di scelta della tipologia di impianti nucleari realizzabili sul territorio nazionale. Tale scelta, importante e complessa per le ovvie implicazioni di sicurezza e di organizzazione, sarà deliberata dal CIPE entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 17 è dedicato all'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Si tratta di una struttura evidentemente fondamentale per la reintroduzione dell'energia nucleare nel nostro Paese. L'esame in Commissione ha prodotto un cospicuo miglioramento delle disposizioni riguardanti tale Agenzia. In particolare, come prescrive l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), è stata esplicitamente disposta, al comma 3, l'indipendenza dell'Agenzia e la sua piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare. Il finanziamento dell'Agenzia verrà effettuato dagli esercenti interessati sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. Signor Presidente, primo luogo, al comma 8 dell'articolo 17 si stabilisce che «sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti». Tale disposizione non appare allineata, collega relatore, con quanto stabilito al comma 6, dove l'Agenzia viene definita «organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri».

Nel complesso, dobbiamo dunque essere grati al Governo Berlusconi per questa coraggiosa innovazione legislativa. È un grande passo avanti sulla via della modernizzazione del nostro Paese. Il centrosinistra, purtroppo, non sarebbe stato mai capace di una scelta così lungimirante.

evidenzia la eterogeneità delle materie ivi trattate che, a mio giudizio, avrebbero dovuto trovare una disamina separata in relazione al contesto di riferimento per una più ampia occasione di dibattito e approfondimento. A ciò si aggiunga che in questo disegno di legge sono contenute ben nove deleghe al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi su temi di non scarso rilievo per il nostro sistema economico, ed in particolare energetico, compreso quello della reintroduzione dell'energia nucleare in Italia. Ma il tutto è coerente con lo stile di questo Governo: affollare le Camere di provvedimenti legislativi che racchiudono i contenuti più disparati, tanto da far mancare spesso il quadro d'insieme complessivo e l'esatta valutazione degli effetti conseguenti e, per la gran parte dei casi, senza apportare contributi di natura strutturale per la crescita del sistema Paese. Nonostante ciò, abbiamo comunque lavorato in Commissione per dare il segno delle nostre proposte ed in alcuni casi il testo del provvedimento è stato modificato anche recependo alcune nostre indicazioni. Vorrei far riferimento innanzitutto ai temi legati all'energia. Quando si interviene con provvedimenti legislativi in materia di energia sono due gli obiettivi principali da perseguire, tra loro assolutamente interdipendenti: da una parte, ridurre i costi dell'energia in generale a carico di famiglie e imprese; dall'altra, creare una nuova strategia economica per uscire dalla recessione, per creare nuovi posti di lavoro e, allo stesso tempo, individuare prospettive di sviluppo nel medio-lungo termine. In ordine al primo aspetto, cioè la necessità che ha il nostro Paese di ridurre i costi dell'energia e quindi migliorare l'offerta equilibrando il *mix* energetico delle fonti, le nostre proposte si sono indirizzate nel senso di integrare le soluzioni delineate dal provvedimento con la promozione del risparmio energetico, della cogenerazione, della generazione di piccola taglia nei pressi dei centri di consumo. Il tutto per consentire maggiore efficienza e più alti rendimenti e quindi aumentare la competitività delle imprese. Ma non possiamo negare che oltre a queste misure, il percorso legislativo serio da intraprendere dovrebbe prevedere norme volte a favorire la concorrenza nei mercati dell'energia, con particolare riferimento al mercato del gas naturale in cui esiste ancora un monopolio di fatto, in cui gli operatori dominanti controllano la gran parte dell'offerta e delle infrastrutture di accesso al mercato italiano tanto da poter dettare sempre e comunque il prezzo imponendolo agli altri concorrenti. Sarebbe arrivato il momento di lavorare per una vera liberalizzazione dei mercati dell'energia, in cui il consumatore sceglie in un contesto di offerta abbondante; ma non lo si potrà fare fino a che non si porterà a compimento un percorso già avviato anche nella scorsa legislatura legislatura di effettiva separazione tra chi controlla la produzione e chi ha il controllo delle reti di distribuzione. Con riguardo al sistema delle imprese, in particolare, si dovrebbero indicare soluzioni e risposte significative per ovviare alle situazioni di assoluto svantaggio rispetto ai *competitors* europei in cui si trovano le nostre piccole e medie imprese. in ragione di un'imposizione fiscale sui consumi energetici che le penalizza a tutti gli effetti senza un'adeguata perequazione. Forse sarebbe opportuno iniziare a pensare a soluzioni volte ad alleggerire i costi di energia a carico di imprese e cittadini, trasferendo il peso degli oneri, per *decommissioning* e rinnovabili ad esempio, dalle bollette alla fiscalità generale. Sotto altro punto di vista, e cioè sul fronte delle prospettive occupazionali e di sviluppo che vengono dal settore dell'energia, il nostro partito in ogni contesto ha sempre evidenziato che una strategia oculata di differenziazione delle fonti di produzione di energia non può prescindere dall'incremento delle fonti rinnovabili. Se esistono alcuni settori in cui le nostre imprese sono leader o comunque lo possono divenire crescendo in ricerca e innovazione, non possiamo farci sfuggire l'occasione di implementare la creazione di vere e proprie filiere nazionali in cui la nostra tecnologia fa da capofila e viene anche esportata. Dobbiamo quindi cercare di creare un sistema di regole certe per lo sviluppo e l'insediamento di queste tecnologie, per agevolare i finanziamenti e gli aiuti pubblici a queste reti di imprese. Tutte le proposte da fare e da noi fatte per il settore energetico hanno risposto e devono comunque rispondere principalmente ad una convinzione di fondo

si deve trasformare in opportunità per il Paese, nel senso del risparmio dei costi dell'energia e della creazione di una nuova frontiera di crescita economica e produttiva che deve vedere i territori come principali attori con politiche e sistemi di incentivazione adeguati. In ordine alle scelte di politica energetica contenute in questo provvedimento, sottolineo come l'introduzione del nucleare ivi prevista richiede comunque tempi lunghi di attuazione ed è lontana dal risolvere le attuali emergenze legate all'approvvigionamento energetico del nostro Paese. Si affida al Governo la delega per l'adozione di conseguenti decreti legislativi che dovranno indicare i criteri da utilizzare per individuare la localizzazione nel territorio italiano degli impianti di produzione dell'energia nucleare e degli impianti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi. abbiamo sottolineato la mancata previsione di una partecipazione adeguata, trattandosi di scelte di rilievo che modificano completamente le politiche energetiche del Paese; abbiamo evidenziato come sia necessario raccogliere il più ampio consenso sociale, creando anche un'adeguata ed obiettiva campagna di informazione. Non riteniamo che la militarizzazione dei siti nucleari quali aree di interesse strategico-nazionale possa considerarsi la soluzione. D'altra parte, abbiamo posto in rilievo quanto fosse inappropriata l'introduzione dell'utilizzo dell'autorizzazione unica senza le procedure VIA (valutazione di impatto ambientale) e VAS (valutazione ambientale strategica). Il tutto con l'intento di porre la massima attenzione sui procedimenti autorizzativi per questi impianti. Non si possono poi non evidenziare altri aspetti critici nell'introduzione del nucleare che vanno vagliati approfonditamente. Voglio far riferimento alla assoluta necessità di coinvolgere l'industria nazionale e il nostro sistema di ricerca, per far sì che l'innovazione in questo settore non venga solo importata dall'estero, e per favorire la riduzione dei costi di realizzazione degli impianti. Che dire ad esempio del fatto che viene demandata al Governo in sostanza la scelta delle tipologie degli impianti di produzione di energia nucleare da realizzare nel territorio nazionale? Vorrei capire a questo proposito se nelle intenzioni del Governo c'è comunque quella di favorire oppure no lo sviluppo di tecnologie e conoscenze tutte italiane nel settore del

per l'alleggerimento dell'*iter* burocratico per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni, grazie alla autocertificazione. Abbiamo dato anche un contributo nella elaborazione

riteniamo comunque condivisibile per raggiungere l'obiettivo di rispondere alla esigenza di repressione di condotte delittuose che stanno sempre più aumentando in questo campo, soprattutto da parte della criminalità organizzata.

quasi all'inizio dell'attuale legislatura. Quando è nato era già vecchio, soprattutto nella parte che riguarda le politiche energetiche e che si può sintetizzare in un'unica idea forte: i problemi energetici dell'Italia si risolvono ricominciando a produrre energia nucleare. Questa da molti mesi è una convinzione ripetuta ossessivamente, in particolare dal ministro Scajola. Forse nel mondo solo il presidente iraniano Ahmadinejad e il mio amico Chicco Testa sono più fissati di lui con il nucleare. Aggiungo che ritornare a parlare concretamente di nucleare poteva essere una cosa utile, la via per sottrarre questo tema alla logica della guerra tra opposte fazioni ideologiche. Ce n'era bisogno e ce n'é bisogno, perché dal referendum del 1987 moltissimo è cambiato anche rispetto al rapporto, tradizionalmente non facile, tra ambiente ed energia: allora il nucleare era visto come la minaccia più grande per l'ambiente; oggi c'è una minaccia, meglio un processo già in atto, ben più temibile e globale come sono i cambiamenti climatici. Oggi ridurre le emissioni che alimentano i cambiamenti del clima, dunque ridurre i consumi di petrolio e di combustibili fossili, è una priorità e un'urgenza assoluta: per l'Italia il nucleare non serve a questo scopo, ma per preparare un futuro senza petrolio è importante che nel mondo, ed anche in Italia, venga intensificata la ricerca per arrivare alla fusione nucleare o a una fissione davvero sicura. La nuova posizione del Governo italiano poteva essere, dunque, la premessa per parlare di nucleare e di energia guardando ai fatti e guardando al futuro; invece mi pare che Governo e maggioranza intendano fare del ritorno al nucleare un tema di propaganda, un altro anello della catena di annunci roboanti e decisionisti, ma generalmente fini a se stessi, che ha segnato questi primi dieci mesi della legislatura. Questa intenzione era già chiara quando è nato il disegno di legge che stiamo discutendo. Un testo nel quale il riduzionismo nucleare cancella i principali nodi da sciogliere per dare all'Italia una politica energetica rinnovata ed efficace: come incentivare l'efficienza energetica, come colmare il *gap* rispetto ai grandi Paesi europei sulle nuove rinnovabili, come spingere la ricerca sulle nuove tecnologie energetiche, dal sequestro dell'anidride carbonica all'idrogeno. È un testo che trascura del tutto i problemi irrisolti del nucleare attuale - le scorie, i costi esorbitanti, i rischi di proliferazione - e propone procedure di tipo quasi militare per scegliere i siti e gestirli, negando ai cittadini l'accesso alle informazioni che riguardano i nuovi impianti. n. 1195 era già vecchio quando è nato, oggi in particolare per la parte che riguarda l'energia, e malgrado alcune modifiche positive introdotte grazie a proposte dell'opposizione (cito per tutte quelle relative all'Agenzia sulla sicurezza nucleare), è decrepito. Dall'agosto 2008 sono infatti successe in Europa e nel mondo cose importanti: nel dicembre scorso l'Unione europea ha approvato il pacchetto di misure sul clima, che non accenna al nucleare e invece fissa obiettivi ambiziosi per migliorare l'efficienza energetica e sviluppare le energie rinnovabili. Da gennaio gli Stati Uniti hanno un nuovo Presidente, che parla pochissimo di nucleare e che invece ha messo al centro dei suoi obiettivi di governo il decollo delle nuove energie ed un programma straordinario per il risparmio energetico nell'edilizia e nei trasporti, di cui è parte integrante la stessa scelta di puntare sulla FIAT come partner di Chrysler. E poi, da alcuni mesi, è arrivata una terribile crisi economica, e tutti i Paesi più grandi ed importanti alla crisi stanno rispondendo puntando sulla cosiddetta *green revolution*. Secondo uno studio recente di HSBC, uno dei principali gruppi bancari del mondo, nell'Unione europea oltre metà delle risorse pubbliche anticrisi sono finalizzate all'innovazione energetica, mentre in Cina la percentuale è del 37 per cento e negli Stati Uniti è di quasi il 15 per cento. Bene, anzi male, perché in Italia solo l'l per cento dei fondi pubblici anticrisi è stato impegnato in questa direzione. Alla base di queste azioni c'è una stessa, ormai generale convinzione: bisogna rinnovare radicalmente il modello energetico nel segno dell'efficienza e delle energie pulite, perché questo impone la crisi climatica e perché questo serve a creare lavoro, a far nascere nuove imprese innovative, ad alleggerire i costi dell'energia per famiglie e per imprese, e dunque serve anche per superare prima e meglio la crisi economica. Come ha detto recentemente Al Gore: «La buona notizia è che le iniziative di grande portata necessarie a porre rimedio alla crisi del clima sono esattamente le stesse che occorre intraprendere per risolvere la crisi economica e la crisi della sicurezza energetica». Il Governo Berlusconi e la sua maggioranza fanno altro, e spesso si muovono in direzione - per dirla con il titolo di un celebre album di Fabrizio De André - ostinata e contraria rispetto al resto del mondo. Ecco un elenco parziale e incompleto dei passi indietro e dei passi falsi accumulati in questi mesi: il tentativo di cancellare gli incentivi del 55 per cento alle ristrutturazioni degli edifici a fini di risparmio energetico, poi fortunatamente rimangiato; il tentativo di boicottare l'accordo europeo sul clima, anch'esso fallito ma che certo non ha giovato all'immagine internazionale del nostro Paese. E poi gli ultimi due episodi avvenuti proprio qui in Senato: il primo, alla vigilia del G8-Ambiente a Siracusa ha messo in imbarazzo persino il ministro Prestigiacomo e il ministro Frattini, costretti a smentire quella ridicola mozione votata in quest'Aula in cui si dice che i cambiamenti climatici non esistono e che se ci fossero produrrebbero più benefici che danni; il secondo riguarda proprio questo disegno di legge: in Commissione industria la maggioranza ha approvato un emendamento del relatore, che cancella il divieto di commercializzare dal prossimo gennaio elettrodomestici bianchi e lampadine a bassa efficienza, una norma che era stata introdotta nell'ultima finanziaria del Governo Prodi e che, oltretutto, comporterebbe un grande vantaggio competitivo per l'industria italiana del settore, all'avanguardia quanto a risparmio energetico. A fronte di tutto questo, resta come sola proposta in positivo il ritorno al nucleare. Si vuole discutere di nucleare? Bene, ma lo si faccia lasciando da parte la propaganda e badando ai fatti. I fatti dicono che nel mondo il nucleare non è certo in crescita. Dicono che costruire una centrale è molto costoso e che per questo le nuove centrali si fanno quasi soltanto in Paesi dove gli investimenti li paga lo Stato. Dicono che da oltre vent'anni negli Stati Uniti non entra in funzione un nuovo impianto. Dicono che se l'Italia realizza 4 centrali da 6.400 megawatt, questo ci costerà non meno di 25-30 miliardi di euro e che il contributo di queste quattro centrali ai consumi di energia sarà inferiore al 5 Dicono che ripartire col nucleare non serve a ridurre la dipendenza dal petrolio (che non viene quasi più utilizzato per produrre elettricità), non serve a fronteggiare la crisi economica, dato che i cantieri non apriranno prima di cinque anni e non serve ad affrontare la crisi climatica, perché i nuovi impianti entrerebbero in funzione dopo il 2020, mentre secondo gli scienziati gli anni decisivi per fermare il *global warming* sono o quindici. Ancora, dicono i fatti che il recente accordo italo-francese, come ha sottolineato tra gli altri un nuclearista convinto come l'amministratore delegato di Ansaldo energia Giuseppe Zampini, conviene solo alla Francia, la cui industria nucleare non trova più sbocchi nel mondo e perciò ha tutto l'interesse a collocare in Italia una tecnologia - quella EPR (*European pressurized reactor*) - già oggi abbastanza vecchia e che fra quindici anni, quando a essere ottimisti entrerebbe in funzione il primo impianto italiano, sarebbe decotta.

tre quarti delle quali sono stoccate da anni in strutture inadeguate in un Comune piemontese, Saluggia, che si trova in un'area idrogeologicamente quanto mai inadatta. E dicono, infine, che nel disegno di legge n. 1195 avete previsto che i siti nucleari verranno localizzati anche contro il parere delle Regioni che li ospitano e che i cantieri nucleari ed i nuovi impianti saranno gestiti come installazioni militari, alla faccia della sbandierata sicurezza intrinseca dei nuovi reattori. La verità è che per affrontare le tre crisi globali nelle quali anche l'Italia è coinvolta - crisi economica, climatica ed energetica - per il nostro Paese il nucleare è un'arma completamente spuntata, ma costosissima, per fabbricare la quale dovremo inevitabilmente rinunciare alle cose più utili, più efficaci, più tempestive. Noi auspichiamo che cominciate a farle queste cose utili, seguendo il cammino dell'Europa e degli Stati Uniti, e che smettiate di baloccarvi e di ingannare il Paese con propositi anacronistici e propagandistici agitati per nascondere il vostro immobilismo. Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, l'economia italiana soffre, ma la sua situazione è meno grave di quella di altre nazioni avanzate; questo è, in estrema sintesi, il quadro emerso dal recente rapporto della Commissione europea. Parto da questo documento perché la sua analisi rivaluta agli occhi del mondo i presupposti su cui si basa il nostro sviluppo, certamente inferiore nel *trend* rispetto alle altre nazioni, ma più solido ed equilibrato. Il merito deve essere attribuito alla propensione al risparmio delle famiglie italiane e alla solidità del nostro settore manifatturiero. Il disegno di legge che stiamo prendendo in esame interviene su alcuni aspetti della vita economica italiana che interessano proprio famiglie e imprese, offrendo strumenti in grado di sostenere questi caratteri peculiari del nostro contesto socio-economico rendendolo più innovativo e competitivo: basti pensare al primo articolo del provvedimento, quello relativo ai distretti produttivi e alle reti d'impresa. Sono ormai alcuni anni che si discute della dimensione delle imprese italiane e della necessità di favorire aggregazione e accordi che le mettano in grado di competere. L'operazione non è così semplice e scontata; non basta superare le naturali resistenze di carattere culturale che gli imprenditori possono manifestare, ma occorre definire nuove regole per giungere ad un sistema di rete che generi reali vantaggi per le singole imprese e allo stesso tempo per l'intero distretto. Il testo del provvedimento va nella giusta direzione, in quanto semplifica i processi di aggregazione e li rende convenienti per le imprese stesse. Altrettanto importanti sono le misure che interessano il turismo. La delega al Governo consente una razionalizzazione e una destinazione mirata degli incentivi a favore di aree territoriali ed enti fieristici che privilegino le zone di eccellenza, evitando una loro distribuzione a pioggia che disperde denaro senza portare risultati apprezzabili. Accanto alla razionalizzazione, un altro aspetto che caratterizza le misure adottate in questo disegno di legge è la semplificazione degli adempimenti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, che credo sia uno dei punti nodali di qualsiasi processo di modernizzazione. Abbiamo infatti un sistema appesantito dalla burocrazia e dobbiamo assolutamente riformarlo se non vogliamo segnare il passo in un contesto mondiale che corre o che comunque ricomincerà a correre. Anche nei percorsi di internazionalizzazione, la delega al Governo, prevista dall'articolo 3-*bis*, di raccolta e coordinamento di tutte le disposizioni legislative in materia, rappresenta una chiave di volta fondamentale ed estremamente attuale per un Paese che sta dimostrando una forte propensione ad inserirsi come protagonista negli assetti e negli equilibri economici mondiali; basti pensare agli accordi che Fiat sta definendo in queste ore. Quanto previsto in questo provvedimento non farà altro che incentivare e rafforzare una naturale tendenza delle nostre imprese ad affacciarsi sui mercati mondiali, accrescendo le loro *chances* di affermazione. Naturalmente, oltre alle dimensioni ed alla giusta organizzazione, per affermarsi nel mondo alle imprese serve presentarsi con prodotti innovativi. Anche da questo punto di vista possiamo contare su una serie di provvedimenti che riordinano il sistema delle aree tecnologiche e delle stazioni sperimentali per l'industria, rendendole più aggiornate e e ammodernate. Sul piano energetico il disegno di legge riesce a definire una visione di interesse nazionale, delegando al Governo una funzione di indirizzo degli interessi statali nel rispetto dei principi del Titolo V della Costituzione libertà d'azione per le Regioni, coerentemente con le esigenze del Paese e con le strategie di sviluppo condivise. In questo quadro si inserisce il tema del nucleare, per il quale il provvedimento delega il Governo ad individuare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, i criteri per la disciplina della localizzazione dei siti, del sistema di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e delle misure compensative da corrispondere alla popolazione. Un aspetto a lungo dibattuto e per anni controverso, quello del nucleare, che oggi trova concorde la maggioranza degli italiani e dei loro rappresentanti in Parlamento. La sua adozione costituisce un cambio epocale non solo dal punto di vista economico ma anche nello stile di vita degli italiani e ambientale. Solo per fare un esempio, prendiamo un Paese vicino a noi, di cui si è parlato poco prima, come la Francia. La Francia produce e utilizza da anni energia nucleare. Nelle case dei francesi i piani di cottura sono piastre elettriche; questo aspetto, che può apparire marginale, marginale, ha invece un grande impatto, sia dal punto di vista della sicurezza che da quello del rilancio economico di molte aziende: basti pensare agli incidenti domestici che avvengono per fughe di gas all'interno delle abitazioni. Molte aziende potranno avviare quindi un processo di innovazione di prodotto, fondamentale per la ripresa e lo sviluppo tecnologico. Non stiamo parlando solamente di energia ma di un'energia pulita a basso prezzo, che sicuramente farà rivedere l'approccio

Sempre in tema energetico l'articolo 18 si propone di disciplinare il mercato del gas naturale per accrescerne l'efficienza e la convenienza. Dare al Governo la delega per la rivisitazione del tetto *antitrust* sulle importazioni di gas, fissato al 2010, è una misura importante perché permette di realizzare dinamiche di mercato virtuose creando le condizioni per un mercato sempre più concorrenziale. Ci sono poi una serie di misure attinenti ai distributori stradali di GPL, che migliorano e rendono più sicuro il sistema distributivo e allo stesso tempo permettono ad un maggior numero di cittadini di usufruire dei vantaggi di questo sistema. Di grande rilievo è anche l'estensione del contributo statale per l'installazione dell'impianto GPL ad ulteriori categorie di vetture. Importanti anche le modifiche della disciplina dei consorzi. Al riguardo occorre sottolineare che i consorzi agrari rappresentano un realtà importante sul mercato agricolo italiano. Ad oggi, secondo l'ASSOCAP, 53 consorzi associati fatturano oltre tre miliardi di euro ed in futuro, secondo valutazioni riportate dalla stampa specialistica, potrebbero rappresentare l'asse portante, insieme con le cooperative, di un piano di rilancio complessivo dell'agricoltura. Ci sono poi altre misure incisive, ma voglio concludere con la *class action* che, adottata superficialmente dal precedente Governo, è stata resa più attuale e al passo con i tempi in questo disegno di legge. Le norme previste per avviare un'azione collettiva sono più agevoli e semplici per i cittadini consumatori, rendendo quindi realmente efficace questo istituto nel momento in cui si voglia farvi ricorso. Quindi, in conclusione, si tratta di un documento molto articolato e vasto che offre al Governo e al Ministero per lo sviluppo economico spazi utili di manovra per accrescere la competitività e per dare slancio a tutto il comparto economico del nostro Paese.

nel 1987 decidemmo l'abbandono della tecnologia nucleare con la paura dei nuvoloni tossici del quarto reattore di Chernobyl, negli occhi di tutti Paesi occidentali. Tutti i Paesi europei ebbero paura, ma noi fummo gli unici a compiere un salto indietro di 30 anni, nascondendo in un cassetto le competenze acquisite. Un Paese moderno, seppur comprensibilmente spaventato, non compie scelte fondamentali per il proprio futuro sulla base di una sensazione, ma fa un'analisi costi-benefici e sceglie il bene della collettività. Una volta presa una decisione, non si ferma davanti al primo corteo dei comitati di paese ed esercita la propria autorità con tutta la forza necessaria e nell'interesse del maggior numero possibile di cittadini. Negli anni Ottanta le condizioni politiche erano differenti e perdere le elezioni poteva ancora significare qualcosa in più di un avvicendamento tra maggioranza e opposizione. Oggi non abbiamo scuse: o siamo in grado di prendere una decisione nell'interesse collettivo e di portarla avanti, nonostante veti e malumori, oppure andiamo a casa e aspettiamo il cambio di governo per dare la colpa a qualcun'altro. Sebbene, infatti, l'Italia abbia spento tutti i suoi impianti nucleari ed i Comuni abbiano fatto a gara a dichiararsi città denuclearizzate, facendo bella mostra di simboletti e bandierine, a meno di 200 chilometri dal nostro confine sono attive ben 13 centrali straniere. Le nubi tossiche si muovono con il vento e possono agevolmente raggiungerci. Quindi, la sicurezza del nostro Paese non è aumentata dopo il *referendum* del 1987 ma è solo stata posta sotto il controllo di Paesi stranieri: alleati ma pur sempre stranieri. cento del nostro fabbisogno viene soddisfatto grazie alle importazioni dall'estero. Che sia gas trasportato via mare, petrolio o energia elettrica prodotta da impianti nucleari francesi poco importa:

perché dovremmo comprare energia dalle centrali atomiche francesi, a due passi dai nostri confini, e non produrla noi? Perché dobbiamo dipendere dai nostri vicini? È stata sufficiente la caduta di un albero in Svizzera per generare il *black out* nella Penisola; in Giappone, nonostante il terremoto di livello otto della scala Richter, le centrali nucleari non hanno smesso, neanche per un secondo, di produrre ed erogare energia elettrica. Quando non cadono gli alberi, dobbiamo sperare che Russia e Ucraina appianino le loro divergenze diplomatiche senza chiudere i rubinetti del gas, per non dover tenere spenti i termosifoni durante l'inverno. Oppure, siamo costretti ad arricchire i produttori dell'OPEC, non tutti proprio ben disposti nei confronti del mondo occidentale e men che mai tolleranti nei confronti del dissenso interno. È un bel paradosso, ma la nostra democrazia, per continuare ad esistere, ha bisogno di appoggiare alcuni tra i Capi di Stato meno democratici del mondo. Diversificare le fonti di approvvigionamento non basterà. Questa strada è stata già tentata, ma le riserve di petrolio sono sempre scarse e concentrate in aree molto lontane dalla nostra influenza. Non lasciamoci ingannare dalle attuali quotazioni del petrolio. Gli analisti concordano nel ritenere che, passata la crisi internazionale (forse già nel 2010), il prezzo del petrolio tornerà a salire consistentemente: probabilmente non fino a raggiungere i 100 dollari al barile ma almeno fino a 70 o 80 dollari. Una seria analisi costi-benefici deve prendere in esame le quotazioni dei prossimi 30 anni, se possibile, per capire la convenienza o meno della costruzione di nuove centrali nucleari. Le energie rinnovabili non sono la soluzione. È necessario che qualcuno lo dica senza ipocrisie. Il sole, il vento e l'acqua sono beni preziosi a nostra disposizione, ma non bastano a tenere accesi i nostri elettrodomestici e in attività le fabbriche. L'orientamento del Governo è di arrivare al 25 per cento di energia elettrica prodotta attraverso le fonti rinnovabili. Mi sembra un obiettivo equilibrato e concreto, anche se l'idroelettrico è già ampiamente sfruttato e l'eolico porta con sé, a mio avviso, una forte controindicazione: deturpa il paesaggio. Siamo sicuri di non preferire una centrale nucleare in una valle, a 1.000 pale eoliche sparpagliate tra i picchi più belli del nostro Paese? Chi sostiene che sia possibile puntare tutto sulle energie rinnovabili dovrebbe anche spiegare agli italiani come consumare un quarto dell'energia che consuma oggi senza rinunciare ad andare a lavorare o a tenere il riscaldamento acceso; oltre al fatto che con l'attuale metodo di produzione di energia elettrica si genera il 27 per cento delle emissioni di CO2 ed il Protocollo di Kyoto prevede salate sanzioni per chi non le limita in tempi rapidi. Bisogna ricordare che fino ad oggi le imprese e i cittadini italiani hanno pagato bollette più care, come minimo del 30 per cento rispetto alla media europea: 11,66 centesimi di euro per 100 chilowattora contro i 7,72 centesimi degli inglesi e i 5 euro dei francesi. I ritardi, i veti, le paure hanno un costo. Per questo apprezzo che nel testo in esame siano indicati la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia, lo snellimento della procedura unica per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di rigassificatori ed il tentativo di contenere l'incidenza dei ricorsi al TAR che hanno sempre fatto lievitare tempi e costi delle grandi opere in Italia. Adesso tocca al Governo localizzare nel territorio nazionale gli impianti di produzione elettrica nucleare e di stoccaggio dei rifiuti radioattivi; non sarà facile. Abbiamo già avuto un assaggio di quanto potrà accadere con le dimostrazioni contro la TAV, il passante di Mestre, il ponte sullo Stretto e lo stoccaggio delle scorie. Dovunque verranno posizionate le centrali, vi saranno proteste; ascoltiamole finché possibile, dopodiché sarà necessario imporre una decisione oppure ripiegare di nuovo con la coda tra le gambe,

È stato un lavoro molto faticoso, un lavoro che ha visto questo provvedimento nascere in un modo, con certe disposizioni, ma quotidianamente

per assecondare sostanzialmente il ritorno al nucleare, ma che in realtà contiene tantissime disposizioni che - mi permetto di dire - sono completamente avulse e stravaganti rispetto al provvedimento nonostante la difficoltà dei lavori che sono stati svolti in Commissione e che quindi rendono anche difficile in sede di discussione generale focalizzare la propria attenzione su alcuni argomenti, essendo tantissimi - lo ripeto - gli argomenti contenuti nel provvedimento, vorrei provare a centrare la mia attenzione e la mia dissertazione su due argomenti che mi stanno particolarmente a cuore, ovvero le politiche energetiche e la *class action*. Per quanto riguarda le politiche energetiche, il Gruppo dell'Italia dei Valori, rappresentato da me in Commissione, ha proposto, attraverso i vari emendamenti presentati, la predisposizione di un piano operativo finalizzato alla promozione della ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento al risparmio, all'efficienza energetica, all'aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile e, soprattutto, allo sviluppo del solare termodinamico, come anche al perfezionamento delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, piuttosto che allo sviluppo del nucleare di nuova generazione a cui, invece, questo provvedimento è improntato.

E quindi, a tal fine, con il disegno di legge al nostro esame intende predisporre procedure autorizzatorie che, in omaggio ad un malinteso principio di semplificazione e celerità, escludono pareri estremamente importanti nella fase predecisoria. il *deficit* di modernizzazione, di innovazione e di efficienza del mercato energetico nel nostro Paese possa essere colmato solo integrando politiche energetiche e climatiche, in un contesto globale in cui sia assicurata la competitività economica e lo sviluppo sostenibile dell'ambiente. Riteniamo, invece, che la posizione del Governo in questo provvedimento sia regressiva. Un Governo che ha lamentato i presunti costi derivanti dall'adesione al pacchetto energetico climatico dell'Unione e che, oltre a rendere più difficile la modernizzazione del sistema produttivo nazionale, penalizzerebbe la ricerca scientifica e le opportunità occupazionali.

e contesta le scelte di fondo che si propone il Governo in carica con questo disegno di legge, perché antistoriche oltre che miopi e solitarie nel panorama internazionale.

ad includere obbligatoriamente nei procedimenti amministrativi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettronucleare, le procedure di VIA valutazione di impatto ambientale - e di VAS - valutazione ambientale strategica - perché solo in questo modo riteniamo si possano rispettare quelle garanzie di sostenibilità ambientale che qualsiasi politica energetica deve portare con sé.

Lo ricordo brevemente: si tratta di un'azione giudiziale di gruppo, dei cui effetti risarcitori possono giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria; tale era stata prevista dal precedente Governo e dall'articolo 140-*bis*

Quindi, uno strumento giuridico utilizzabile - lo ripeto - da soggetti collettivi per garantire la tutela di interessi collettivi, tanto che le associazioni dei consumatori e gli altri soggetti rappresentativi degli interessi collettivi, portando in giudizio e facendo portando in giudizio e facendo condannare imprese o pubbliche amministrazioni che abbiano provocato un danno ai singoli, permetterebbero ai singoli stessi, che in forza della sentenza di condanna ne avessero i requisiti, di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno. secondo il testo che oggi è stato approvato, la *class action* corrisponde semplicemente alla possibilità per un soggetto di associarsi ad un altro soggetto al fine di tutelare un identico diritto individuale. Come capite, c'è una grossa differenza. Legittimato oggi ad esperire la *class action* è dunque ciascun singolo - ed eventualmente solo un soggetto collettivo - e il diritto al risarcimento del danno è riconosciuto solo a chi abbia avviato la *class action* e a coloro che, entro un termine perentorio, abbiano presentato un formale atto di adesione alla stessa. È evidente che, con tale modifica, vi è un intento deflattivo rispetto all'esercizio di questa azione. Un altro elemento che per noi era fondamentale - e che ritorna in Aula attraverso un nostro emendamento - è il fatto che nel testo proposto dal Governo si parla solo di atti illeciti di tipo contrattuale e non quindi anche di atti illeciti di natura extracontrattuale. Anche da questo punto di vista è evidente, soprattutto per per i giuristi, che c'è una grandissima differenza rispetto all'onere della prova e rispetto ai termini di prescrizione. Riconoscendo una tutela all'illecito contrattuale ed extracontrattuale si arriverebbe ad una tutela maggiore del consumatore. Invece, anche in questo caso, la proposta del Governo - che non è più una proposta, ma è una cosa concreta - va esattamente nella direzione opposta. Concludo, signor Presidente, ricordando un altro elemento che, come giurista, mi sta particolarmente a cuore. In questo provvedimento è stata approvata un'altra norma che io ritengo aberrante dal punto di vista giuridico. Si è voluto infatti concentrare davanti al tribunale amministrativo del Lazio, prevedendo quindi una competenza territoriale e una giurisdizione territoriale esclusiva,

in sede di discussione su questo provvedimento perché esso contiene, agli articoli 14 e 15, una delega al Governo in materia di energia nucleare e di localizzazione dei siti per la produzione di energia elettronucleare, argomento sul quale, fin dalla XIV legislatura, ho presentato disegni di legge che, con questo provvedimento in discussione, per iniziativa del Governo diventeranno legge dello Stato. Il nucleare è oggi la primaria fonte di energia, alla quale accedono anche Nazioni produttrici di altre fonti primarie (quali petrolio, gas naturale e carbone) e a cui hanno diritto anche Nazioni in via di sviluppo. La cooperazione per l'uso pacifico del nucleare è indispensabile per garantire a tutti l'uso dell'atomo, ma, al contempo, si debbono evitare i rischi di proliferazione. L'uso del nucleare è necessario per diminuire la dipendenza globale dal greggio, a dispetto di una domanda di energia in aumento dappertutto, compreso il cosiddetto Terzo mondo e per favorire lo sviluppo di una forma di energia che non inquina. l'indipendenza dal petrolio raffredda anche le tensioni che hanno caratterizzato il secolo scorso e che sono comunque presenti nell'area del Medio Oriente e delle guerre che l'hanno insanguinato. Il ciclo energetico del terzo millennio è sicuramente fondato sul nucleare, così come nell'Ottocento lo era sul carbone e nel Novecento sul petrolio e sul gas naturale. Il passaggio dal petrolio e dal gas naturale al nucleare sarà ancora lento, tuttavia l'uso di reattori sempre più sicuri e la possibilità di riuscire in tempi brevi a riciclare le scorie imporrà sicuramente una significativa accelerazione in favore di questa fonte di energia. Sul piano dei rapporti internazionali, la geografia del nucleare apre nuove prospettive perché russi e americani si propongono due obiettivi fra essi compatibili. Da una parte, la Russia offre lo sterminato entroterra del suo continente alla costruzione di nuove centrali ed al deposito delle scorie, mentre gli Stati Uniti e l'Occidente si impegnano nella ricerca per la costruzione dei reattori cosiddetti autofertilizzanti. Davanti a questa prospettiva non può l'Italia esprimersi affidandosi fideisticamente alle fonti alternative e ai distributori di combustibili fossili. È imperativo un ritorno dell'Italia al nucleare. L'idea che qualcuno alimenta del ritardo della nostra Patria nella tecnologia dell'atomo non è un buon alibi per non impegnarci nella ricerca e nella costruzione dei reattori atomici. Per questo i disegni di legge

da una *impasse* che è durata troppo tempo, oltre vent'anni, e consentono così all'Italia di ritornare, unica Nazione oggi fra i G8 esclusa dalla produzione di energia elettronucleare, fra i Paesi che possono accedere anche a questa fonte di energia, così come avviene per gli altri Paesi del G8. La Francia produce l'80 per cento della sua elettricità con il nucleare, ma anche Nazioni come Slovacchia e Ungheria raggiungono cifre significative con circa il 65 per cento. La tanto ammirata Europa progressista ha fatto del nucleare un pilastro della propria politica energetica. La Germania, additata sovente come una delle Nazioni che di più si è impegnata nella ricerca delle fonti energetiche alternative, ricava dall'atomo il 31 per cento della sua energia, la Spagna il 26 per cento ed il Regno Unito il 22 La Gran Bretagna ha inoltre programmato di costruire sei nuove centrali. In Europa operano 164 reattori nucleari, con una produzione che sfiora il 30 per cento dell'intera energia elettrica del continente. Il punto essenziale è però quello delle prospettive future. La domanda di energia, ovvero i consumi, cresce esponenzialmente e la risposta non può essere affidata fideisticamente - lo dicevo prima - alle energie alternative o ai combustibili fossili, i cui giacimenti non siamo certi di stimare, e che sono politicamente causa di instabilità. Si pensi a come è stato trattato il Medio Oriente. Esso è stato considerato una regione della quale, finché avesse continuato a pompare petrolio, nessuno avrebbe avuto interesse a mutarne le condizioni politiche e sociali. Oggi è tutto cambiato e la sicurezza dei nostri Stati passa anche nella maggiore autosufficienza energetica. Non possiamo tuttavia affidarci alle energie alternative perché il loro contributo alla richiesta di elettricità è modesto e difficilmente espandibile. Per produrre 1.000 megawatt sarebbero necessari 17 chilometri quadrati di pannelli fotovoltaici, difficili da installare nei nostri territori fortemente antropizzati. Ma 1.000 megawatt sono la produzione di energia di un normale reattore. Ciò che è urgente è la capacità di risposta ai fabbisogni e l'energia nucleare è la più rapida da produrre, ma anche la più concorrenziale in termini economici. Con il petrolio ed il gas soggetti a continue speculazioni, gli stessi estrattori di tali materie prime hanno continuato a sviluppare il nucleare, e ciò vale in particolare per gli Stati Uniti e il Regno Unito, ma anche per tutti gli altri produttori di combustibili fossili. Poiché la produzione di energia è il vero potere economico dei Paesi industrializzati, l'Asia (peraltro povera di petrolio e gas) ha avviato una sistematica costruzione di centrali. La Russia è talmente consapevole di ciò da ipotizzare un ritorno al ruolo di superpotenza proprio grazie alle sue enormi riserve di fonti di energia primaria, *in primis* il gas, che è sei volte superiore a quello degli altri Paesi europei, senza tralasciare, tuttavia, un forte e crescente impegno nel nucleare. Con buona probabilità, entro il 2015 Mosca sarà in grado di determinare direttamente i prezzi dell'energia. Mosca pensa a un rilancio del nucleare con l'obiettivo, per il 2020, di produrre energia tramite il nucleare per almeno il 25 per cento (ora è al 14 per cento). Vorrei altresì ricordare che la nostra Europa politica è nata con la Comunità europea dell'energia atomica il suo padre fondatore, Jean Monnet, affermò che l'energia atomica è l'essenza della politica di potenza nazionale. Vi è inoltre una questione etica, oltre che economica e politica, per chi si oppone alla costruzione di centrali nucleari nel nostro Paese. L'ENEL ha acquisito la Slovenske Elektrorbe, primo operatore slovacco e possessore di sei reattori che nel 2003 hanno contribuito per il 69 per cento alla produzione di elettricità della Slovacchia.

del G8, in particolare Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Russia, allo sviluppo dell'energia nucleare. Ciò che qualcuno non vuole per la nostra Nazione, ossia l'energia nucleare, è però dal medesimo considerato una buona cosa se prodotta al di fuori dei confini nazionali; non solo, è anche indicato come un affare sotto il profilo economico, poiché l'impegno di spesa sarà ampiamente remunerato nel corso degli anni dal minore costo della produzione elettrica e dall'inferiore dipendenza italiana dai produttori di combustibili fossili. Nonostante l'Italia non abbia sul suo territorio centrali nucleari, essa partecipa, come abbiamo visto, alla produzione di energia elettrica con l'atomo. Ciò dovrebbe anche far venire meno le ragioni di chi sostiene che, non avendo noi sviluppato tale sistema, non abbiamo più le valenze tecniche e le conoscenze scientifiche per iniziare tale processo produttivo. Ciò non è vero, perché ho appena ricordato come l'Italia partecipi attivamente allo sviluppo dell'attività nucleare in molti altri Paesi. altri Paesi. Allo stato attuale l'Italia è costretta ad acquisire energia elettrica dall'estero con grande guadagno per gli esportatori, essendo il costo dell'energia in Italia di gran lunga il più alto in Europa, con oltre 100 euro/Mwh, contro i 55 euro/Mwh del centro Europa, dove vi è abbondanza di impianti nucleari e carbone, da noi assenti o poco impiegati. intervento con un piccolo conto, ma esemplificativo. In Italia i consumi di energia elettrica sono stati nel 2005 pari a 330.000 Gwh. Se si confrontano i costi tra la media europea e il costo italiano, si ottiene un numero spaventosamente grande:

ossia una finanziaria all'anno, che noi dilapidiamo nel sovrapprezzo dell'energia. Ogni anno bruciamo quindi il valore di una manovra

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa maggioranza ci ha ormai abituato a provvedimenti disorganici, confusi, spesso superficiali e contraddittori. È un metodo che nasconde un sostanziale disinteresse verso l'attività legislativa e, come tale, cozza con lo spirito, oltre che con la sostanza, della Costituzione.

È quasi un anno che circola nelle Aule del Parlamento dalle quali esce profondamente mutato e, pur tuttavia, sempre disarticolato e caotico con un insieme di articoli che mettono insieme materie di tutti i tipi: dai consorzi agrari, alla contraffazione, fino alla ripresa della produzione dell'energia nucleare nel nostro Paese. aspetto che mi sta particolarmente a cuore perché, pur non avendo pregiudizi sull'uso dell'energia nucleare, faccio fatica a vedere come la maggioranza cerchi di far ripartire un'avventura interrotta nel 1987 per volontà popolare con un *referendum* e lo fa con una pesante eredità, quella delle scorie, tuttora irrisolta. Quando questo disegno di legge approdò alla Camera dei deputati suscitò già allora preoccupazione e stupore nelle file dell'opposizione e nell'opinione pubblica il fatto che il Governo proponeva di riprendere l'installazione di centrali nucleari con una norma che si limitava a delegare questo ribaltamento di prospettiva a due articoli che, in sostanza, prevedevano che il nucleare era un affare del Governo e che Regioni ed enti locali non c'entravano, che la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate potevano essere materie di una succinta delega al Governo. Anche il Parlamento era del tutto fuori da ogni possibilità di controllo, insieme alle Regioni e agli enti locali, come se si immaginasse davvero un Paese nel quale era possibile installare una centrale nucleare decidendolo *manu militari* con il Governo, seduto magari ad un tavolo apparecchiato per le sole imprese costruttrici. Una delibera CIPE doveva definire le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che potevano essere realizzati nel territorio nazionale senza nessun serio impegno sulla sicurezza, sullo stoccaggio delle scorie, sul *decommissioning* delle vecchie centrali a fine vita. Un problema tutt'oggi irrisolto e che la dice lunga sui tempi della nostra amministrazione in materia di nucleare. Il provvedimento, per fortuna, è uscito dalla Camera, grazie a una battaglia serrata del Partito Democratico e delle altre opposizioni, che era già tutta un'altra cosa. Recava varie misure volte a garantire la sicurezza e il potenziamento del settore energetico, istituiva - soprattutto - l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare che, come ha precisato successivamente il Senato, secondo la normativa europea deve essere indipendente ed operare in piena autonomia, imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, irrogare sanzioni amministrative, disporre la sospensione delle attività e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. L'Agenzia ha dunque il compito di garantire la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale ma è sempre, ahimè, di nomina governativa. Il Senato ha precisato molti altri aspetti: la concomitanza tra la disciplina per la localizzazione della produzione di energia elettrica nucleare e quella dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi; il riconoscimento di benefici non solo alle persone residenti e alle imprese, ma anche agli enti locali; il fatto che l'autorizzazione unica non sostituisca le procedure di VIA e VAS, cui si deve obbligatoriamente ottemperare; la previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali; la costituzione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e delle opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia. Dunque, il provvedimento che stiamo discutendo chiarisce meglio una serie di questioni, ma ciò non è sufficiente per farci dire che siamo tranquilli sullo sviluppo della produzione di energia nucleare nel nostro Paese. Un Paese dove, come si è visto in Abruzzo, è possibile ancora costruire senza le regole elementari della sicurezza. Gli italiani hanno votato no al *referendum* non solo per l'impatto che ebbe la vicenda di Chernobyl quanto anche per l'impatto delle notizie provenienti da casa nostra, soprattutto per quanto riguarda le centrali di Trino Vercellese e quella di Borgo Sabotino, vicino Si dirà che molta acqua è passata sotto i ponti da quel *referendum* abrogativo che nel 1987 cancellò in Italia per molti anni la prospettiva di una ripresa della produzione di energia nucleare. Molti sostengono che ora le cose sono diverse, che siamo alle centrali di terza generazione o di terza generazione e mezza, ma queste centrali per quanto più sicure delle precedenti non risolvono il grave problema delle scorie. Quindi, che cosa è cambiato che possa far cambiare quell'orientamento imposto dai cittadini italiani a larghissima maggioranza? La paura determinata dalla crisi petrolifera, il fatto che in Italia si è fatto ben poco in tema di risparmio energetico e di sviluppo di fonti alternative. Rimane comunque la domanda: prima di arrivare ad avere un significativo apporto di energia dal nucleare quanti anni passeranno? Almeno un decennio, se si vuole credere ai più ottimisti. Non sarebbe meglio aspettare le centrali di quarta generazione, che sembrano risolvere buona parte dei problemi del vecchio nucleare? In questi giorni l'Italia è al centro dell'attenzione del mondo per l'accordo FIAT-Chrysler. Quell'accordo si fonda su una tecnologia che sposa efficienza e concezione ecologica dello sviluppo. Oggi non esiste ancora una tecnologia in grado di eliminare il problema dei problemi, quello delle scorie, quindi il nucleare è fattibile solo se, in concomitanza con l'individuazione dei siti dove allocare le centrali, si individueranno anche i siti per lo stoccaggio delle scorie. Diciamolo chiaramente, quanto tempo ci vorrà? Mettiamo che si parta domani mattina e si decida che in un determinato luogo, in una qualche Regione, si collocheranno centrali nucleari. Che cosa si farà per convincere la popolazione? Non bastano i sondaggi, ammesso che siano veri,

cosa si farà ? Si manderà l'esercito come a Napoli? D'altronde, per convincere la gente ci vorrà molto tempo. Chiunque abbia un minimo di buon senso sa che oggi il costo dell'energia nucleare è inferiore solo se al costo della produzione pura e semplice non si unisce quello dello stoccaggio e quello della messa in sicurezza dei siti, del trasporto delle scorie nucleari e del *decommissioning* a fine vita. Per non parlare dei costi ambientali che nessuno è in grado di quantificare e che stiamo buttando sulle spalle dei nostri pronipoti. Stiamo andando in controtendenza anche perché non abbiamo sviluppato le energie alternative

Non c'è chi non veda, al di là delle comodità dei nostri Palazzi, che all'esterno vi è un Paese che arranca, un Paese che si muove con difficoltà rispetto al resto del mondo, un Paese che ha raggiunto livelli di progresso e di benessere che

In questo provvedimento, il nostro grande ministro Scajola (e mi piace così qualificarlo) ha pensato, con impegno e competenza, di enunciare (perché di un'enunciazione si tratta), affidandosi al Parlamento, tutto ciò di cui il nostro Paese abbisogna per tornare ad essere una delle prime potenze industrializzate del mondo e per non correre il rischio di andare verso la coda dei sistemi produttivi di avanguardia nel mondo. Sono allora previste la riforma degli interventi per la reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca e sviluppo ed altre forme di incentivi. Sappiamo bene che cosa significa perdere enormi sacche di occupazione: si pensi per un momento al settore tessile, abbigliamento e calzaturiero in Puglia, all'industria degli occhiali del Nord-Est, a tutte le attività manifatturiere ed a tutte quelle attività di impresa nelle quali il costo del lavoro e la componente personale la facevano da padrone. padrone. Posto che noi in questo ambito non possiamo più operare per essere sufficientemente competitivi come lo eravamo una volta, bisogna pensare a conseguire economie serie,

la volumetria degli immobili in Italia del 20 per cento senza passare dai Comuni, ha avuto tanto successo ed è stato così favorevolmente accolto? La risposta è presto data: il cittadino il cittadino italiano non riesce più a sopportare le involontarie angherie che la pubblica amministrazione, la pur benemerita burocrazia, non riesce più ad affrontare e risolvere. allora il problema dei problemi: l'ammodernamento dello Stato, l'ammodernamento del sistema produttivo e l'evoluzione del suo apparato in chiave utilitaristica (o, come detto, di reindustrializzazione), l'attenzione notevole alla ricerca ed allo sviluppo e quindi ad altre forme di incentivi (che non fossero quelli che in passato ci hanno consentito di realizzare gli insediamenti produttivi - perché no - anche la grande e notevole occupazione che fece di questo Paese la quinta potenza industrializzata del mondo), l'attenzione ai consorzi agrari, ambito al quale noi siamo oltremodo ossequiosi. Chi conosce bene la legislazione in materia sa che questa fu ritenuta la più grande opera di ingegneria societaria mai inventata al mondo, ma per un lungo periodo, dacché entrarono in crisi a motivo della loro burocratizzazione, abbiamo dovuto subire il linciaggio di questo grande istituto, che merita di essere rivitalizzato. Ancora oggi esistono, infatti, in Italia i problemi propri della polverizzazione del settore agrario, che nessuna soluzione, nemmeno la cooperazione di primo, di secondo e di terzo livello, pur sussidiata e finanziata al 100 per cento dallo Stato negli anni decorsi, ha consentito di risolvere. Ecco allora il rilancio dei consorzi agrari, l'internazionalizzazione delle imprese.

per la pianta che si piega al passare del vento, ma, ahimè, non riesce ad avere la struttura necessaria per poter competere in un mondo globalizzato sotto il profilo economico. Ecco, allora, la SIMEST, un istituto virtuoso, una società a capitale pubblico che ha dato tanta soddisfazione laddove è stata applicata; chi l'ha conosciuta ed ha visto come ha lavorato nei Paesi dell'Est europeo, nello sviluppo della nuova Europa, può certamente apprezzare l'attenzione che il Ministro rivolge a tale società e anche all'utilizzazione dei suoi frutti nella logica del potenziamento e della capitalizzazione delle imprese dell'Est europeo. tutela finale dei diritti di proprietà industriale, vorrei ricordare quante volte un'inadeguatezza della legislazione in materia ha fatto sì che chi ha inventato il prodotto ed è riuscito a diffondere il *made in Italy* nel mondo ha dovuto subire la concorrenza sleale e a volte ricomprare i marchi che qualcun'altro con una legislazione più forte ha potuto registrare altrove, pur essendo stato un frutto dell'ingegno italiano. Quanto alla delega al Governo in materia nucleare, chi di noi non vorrebbe soluzioni che non implicassero preoccupazioni, ma è evidente che la stagione è così particolare che la globalizzazione del sistema produttivo insieme all'impossibilità di fermare alla frontiera l'eventuale rischio del nucleare ci mettono nelle condizioni di dire che non possiamo restare fermi. Chi, come noi, sa quant'è lunga l'Italia l'Italia ed è stato contattato dalle imprese che continuano a lamentare l'impossibilità di competere con il resto del mondo perché il costo energetico, che rappresenta non meno del dieci per cento del costo in Italia arriva almeno al 30 per cento in più, non può non rendersi conto che nessun corridore, nemmeno Zatopek, può vincere la corsa, se qualcuno corre molto di più e a condizioni molto più agevoli.

gli ambiti del nuovo sviluppo ai fini della produzione di energia, che non sarà solo nucleare, perché nel provvedimento, onorevole ministro Scajola, si parla anche di impianti eolici, nonché dell'ammodernamento della rete distributiva per il gas metano.

con la collaborazione e la condivisione delle forze che oggi non sono al Governo e che sono altrettanto virtuose nell'impegnarsi, vi invito ad andare avanti perché in quest'Aula, dagli interventi che si sono succeduti fino a questo momento, ho ravvisato

Signor Presidente, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, è in discussione un provvedimento che giunge in Aula per l'esame dopo un impegnativo *iter* in Commissione. Commissione, diverse componenti hanno condiviso le perplessità da noi evidenziate ma purtroppo la logica dei numeri e la pressione del Governo hanno impedito modifiche sostanziali al disegno di legge. Il provvedimento nasceva per finalizzare un efficace riordino organizzativo e di larghe prospettive per il sistema industriale del Paese ma, per esigenze di *marketing* politico legato a vicende che precedevano la crisi quando ancora il prezzo del petrolio era alle stelle, è diventato lo strumento cui viene affidata una *mission* istituzionale per reintrodurre il tema dell'energia nucleare, tema non all'ordine del giorno alla luce delle risultanze del *referendum*. A nostro avviso sarebbe stato più opportuno elaborare un apposito provvedimento che tenesse conto degli strumenti istituzionali, dei collegamenti con i territori e dei rapporti con i cittadini che sono stati bypassati da sondaggi a campione. Un rullo compressore che ha deviato il percorso originario che dava il titolo al provvedimento, scavalcato da un semplice «nonché in materia In queste ultime legislature non ho mai visto tanti emendamenti presentati in Commissione dall'Esecutivo, a seguito di scelte che meriterebbero impegni di spesa che però il Governo non è in grado di garantire.

che, riconosciuti come abitanti del Paese del sole, produciamo meno energia solare addirittura della Germania. Quando presentiamo questi argomenti non andiamo come voi alla ricerca di vantaggi mediatico-elettorali. Vogliamo configurare una Nazione in cui il consenso sociale non si basi sull'approssimazione, ma si fondi su risultanze più concrete e durature che diano sicurezza e non danneggino la salute delle generazioni future. Questa è la vera *mission*:

Esistono inventori, scienziati, aziende che hanno in mano buone soluzioni che però non sono sostenute doverosamente dalla politica. Creiamo un luogo di incontro per presentare progetti concreti che diano risultati in poco tempio e garantiscano l'ambiente, senza trincerarsi nel non fare perché sarebbe meglio

l'Esecutivo, che porta a casa il federalismo fiscale utilizza invece i FAS, che sono risorse finanziarie addizionali, come un vero proprio bancomat che con l'aiuto al Mezzogiorno non c'entra nulla. Infatti, il Governo ricorre ai FAS anche per ripianare i disavanzi di spesa corrente degli enti locali. Oggi, paradossalmente, è possibile dire che con i fondi destinati al Mezzogiorno si aiuta tutto il Paese, dimenticando che per regolamento il FAS ha un carattere addizionale ed è un fondo aggiuntivo e straordinario. A questo punto permettetemi una digressione da meridionale e da siciliano. Il vero *coup de théâtre* lo abbiamo registrato ieri, proprio al teatro Massimo al teatro Massimo di Palermo dove il ministro Scajola e il sottosegretario Miccichè, emulo di "papi" Silvio politico, come se fossero a «Porta a Porta» (senza Vespa, però), hanno firmato davanti ad un notaio un contratto con gli impegni che il Governo intende mantenere nel corso di questa legislatura. FAS dovevano arrivare ieri, non tra quattro anni. Si rimane di ghiaccio ascoltando il ministro Scajola che vuole trasformare il Sud in un volano per l'economia nazionale, dai fondi europei, alle zone franche urbane, agli aiuti alle imprese. Dove sono i venti miliardi scippati alle risorse del Mezzogiorno? Perché non restituiscono i quattro miliardi dei Fas spettanti alla Sicilia? Perché non reinseriscono il credito di imposta voluto e promesso alle imprese? A proposito di imprese, ho ascoltato alcuni numeri: 150.000 imprese hanno aperto la partita IVA; 200.000, invece, hanno chiuso i battenti. È questa la verità. La verità del colpo di teatro sta nel fatto che il Sottosegretario ha dichiarato che in Sicilia abbiamo spazi infiniti per il nucleare. Io chiedo: anche per le scorie? La Sicilia, caro Miccichè, ha già dato. Basta guardare alle percentuali di tumori e di morti a Gela e a Priolo. Basta con i ruffiani del re! Restituite alla Sicilia ed al Sud il maltolto! Per tornare al merito del provvedimento, io ritengo che dobbiamo puntare con più energia ai temi riguardanti i distretti industriali e le reti d'impresa. e le reti d'impresa. Nell'immaginario collettivo, purtroppo, si è ingenerata l'idea che l'internazionalizzazione delle imprese sia un sinonimo di risparmio sui costi del lavoro: fabbrico all'Est e vendo in Italia, ma con danni irreversibili all'occupazione. Internazionalizzazione delle imprese significa, invece, cercare nuovi mercati fuori dall'Italia per proporre la qualità del nostro prodotto. Il percorso che la FIAT sta attuando ci aiuta a comprendere meglio il concetto. Su questo argomento, in Commissione abbiamo detto la nostra, così come Abbiamo svolto un buon lavoro, confortati anche dall'audizione con i rappresentati delle categorie produttive, e mi auguro che gli emendamenti presentati abbiano, così come quello sulla piccola editoria, maggior fortuna a vantaggio dello sviluppo economico ed occupazionale dell'intero Paese. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un provvedimento molto vasto, che interviene in molti settori e contiene misure importanti al fine di determinare di determinare maggiore concorrenzialità e apertura del mercato e di dare un'iniezione di competitività alle aziende italiane. La prima parte dell'articolato prevede, infatti, una delega al Governo per disciplinare la configurazione giuridica delle reti d'impresa. Auspico che il Governo realizzi l'obiettivo dichiarato dichiarato di semplificare le norme, agevolando l'accesso al credito, specialmente per le piccole e medie imprese, e riducendo gli oneri per le stesse. Infatti, il sistema produttivo non può essere rilanciato senza riordinare quegli organismi che affollano il quadro operativo e senza semplificare le norme e le procedure. Mi trova d'accordo l'attenzione che il provvedimento pone sullo sviluppo delle nuove tecnologie e sulla ricerca innovativa. Per quanto concerne lo sviluppo del commercio internazionale e gli interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese, è importante riordinare gli enti e gli istituti del settore al fine di renderli più funzionali. Tuttavia, ciò non basta. Il provvedimento contiene, altresì, misure importanti per combattere la contraffazione, nonché misure a favore

Con nostro rammarico, è stata eliminata la possibilità di avviare cause collettive da parte dei cittadini coinvolti nei grandi crack finanziari del passato (ovviamente, penso ai casi Parmalat e Cirio). Reputo, invece, positive le misure sull'utilizzo di immobili militari per l'installazione di impianti energetici e approfitto per sollecitare il Governo a potenziare e favorire lo sviluppo di centrali idroelettriche, che sappiamo essere sicuramente più rispettose dell'ambiente rispetto alle centrali nucleari.

Io ho ascoltato lei, non la sto provocando; lei ha provocato gli altri perché non ha parlato della legge. Di fatto lei della legge non può parlare male per il semplice motivo che è uno dei tanti che nella scorsa legislatura andava dicendo che avreste realizzato esattamente quello che stiamo realizzando noi, tolta l'energia nucleare, che non vede lei tra i maggiori proponenti; ma sa benissimo, provenendo dalla Sicilia, che ormai sono cambiate le cose dal 1987. Oggi vada a dire ai suoi

Pertanto, chiedo scusa, ma spero che domani, nel corso dell'esame del provvedimento, siate coerenti almeno con quanto avete detto in questi anni. Ci avete detto che nella scorsa legislatura non potevate fare niente a seguito delle pressioni dei Verdi e degli altri piccoli partiti; oggi che non ci sono,

qualsiasi cittadino, e che anche voi avreste dovuto fare, cioè cercare di riammodernare il sistema Italia soprattutto per quanto riguarda l'energia. Sapete benissimo che le industrie più fiorenti dell'Italia sono energivore, quindi non possono essere concorrenziali se non hanno il giusto costo. Pertanto, tutti,

ha partecipato, senza naturalmente avere la possibilità - com'è ovvio - di stravolgerlo, c'è stato un netto miglioramento. Su questo mi vorrei soffermare per non ripetere le cose che hanno detto in tanti, in particolare su due argomenti che l'opposizione non ha toccato, uno dei quali riguarda la contraffazione. Voi sapete benissimo che una delle industrie più importanti della nostra Nazione è l'idea, è la fantasia, è soprattutto il piccolo artigianato; quel piccolo artigianato che ha permesso alle industrie di produzione di pelletterie ed altro di portare ricchezza all'Italia. GARRAFFA *(PD)*.

io non l'ho interrotta, l'ho ascoltata, gentilmente. Se lei mi ascolta, probabilmente imparerà qualcosa, almeno per potermi criticare, ma su fatti concreti. Sulla contraffazione lei ha avuto modo di dire che voi avete fatto delle modifiche. Mi trova d'accordo: siete stati voi, ben venga; la legge la stiamo facendo anche in materia di contraffazione, che è un argomento interessante.

si usa materiale radioattivo, che produce scorie. Quindi, anche per scopi estremamente importanti, noi già produciamo delle scorie radioattive e abbiamo delle centrali bloccate, che continuano a perdere danaro, perchè dobbiamo mantenerle in sicurezza.

Chiedo scusa al Presidente, forse la tarda ora ci porta a scherzare e, forse, a trascendere. Rimane il fatto, comunque, che questo provvedimento, al di là delle valutazioni dell'Aula, è stato recepito dalla gente come un atto veramente importante. C'è una grande speranza, una grande aspettativa; il lavoro non si crea senza dare strumenti. Abbiamo parlato della contraffazione, qualcosa che in gran parte degli interventi è stato dimenticato.

anche nelle scorse legislature perché - ripeto - il problema del costo dell'energia era ed è un qualcosa che è impossibile non affrontare. Pertanto, mi auguro

nel frattempo ha dovuto accogliere, come è stato ricordato, molte integrazioni e molte modifiche. Questo naturalmente perché dalla elaborazione della manovra finanziaria ad oggi lo scenario economico è così profondamente mutato da richiedere un'azione sempre più incisiva per combattere una crisi tra le più gravi che la storia dell'economia industriale ricordi. Quindi, è un po' difficile intervenire a commento di un provvedimento estremamente articolato, che copre argomenti che vanno dall'energia ai trasporti, dai distretti industriali alle reti di impresa, fino agli incentivi al commercio estero. Tuttavia, ci tenevo a farlo perché c'è, in qualche modo, un filo conduttore che unisce quasi tutte le misure del provvedimento e, credo, al tempo stesso costituisce una chiave di lettura da parte del Governo di questa crisi che stiamo attraversando e degli strumenti con i quali possiamo farvi Una crisi che si radica nell'eccezionale squilibrio tra un blocco di Paesi gravitante sulla Cina, che ha fatto il suo ingresso nell'economia globale monopolizzando la produzione manifatturiera a basso costo, e un blocco di Paesi gravitante intorno agli Stati Uniti, che ha continuato ad espandere i propri consumi pur avendo perso gran parte della produzione e finanziando gli acquisti con un crescente ricorso all'indebitamento. Naturalmente si sono moltiplicati gli strumenti di credito, che sono stati, quindi, di qualità via via più scadente, e il sistema creditizio ha mirato a disfarsene, ribaltandone il rischio sui risparmiatori. La crisi del sistema bancario, diffusa, generando la contrazione del credito, e il virus finanziario si è trasferito all'economia reale. Dunque, una crisi strutturale che era, in fondo, largamente prevedibile, per la verità largamente prevista dalla letteratura economica anche se gran parte di questa è ignorata dai *media* dai *media* e dalla classe politica. Ebbene, rispetto a tale crisi è davvero un luogo comune sostenere, come tanti fanno, che dato che l'economia è globalizzata, se ne entra insieme e se ne esce insieme. Non è così. Ne esce meglio e prima chi è riuscito a cogliere l'occasione della crisi per compiere la transizione e la trasformazione necessaria. Ne esce meglio e prima chi è riuscito a recuperare produttività e competitività nel momento della crisi.

auspicato e molto caldeggiato dalle tendenze neostataliste (che forse nascondono il desiderio della politica di rimpossessarsi dell'economia e del mercato), ma, al contrario, attraverso aiuti alla produttività e alla competitività del sistema produttivo, in cui le imprese private devono continuare a confrontarsi, in un contesto di mercato e di concorrenza che è l'unico che favorisce l'innovazione e l'efficienza. Credo che sia sbagliato addossare le colpe di questa crisi al mercato e al liberismo. Credo, al contrario, che le misure di questo decreto, puntando proprio a ristrutturare la competitività e la produttività del nostro sistema economico, economico, comincino a percorrere la strada giusta e rappresentino un tassello importante nella strategia del Governo. Queste misure, che sostengono la produttività del sistema nel medio e nel lungo periodo, non sono contenute solo in questo pensiamo alle misure che riguardano il settore dei trasporti e delle relative infrastrutture; pensiamo alla riforma dell'istruzione universitaria, che serve ad elevare la qualità della formazione; pensiamo alla riforma della macchina pubblica e della pubblica amministrazione, tesa a dare maggiore efficienza al sistema dei servizi pubblici - però certamente anche

la piccola impresa si crea le condizioni per diventare grande o se ci sono le condizioni per sfruttare le economie di rete e le economie esterne, che si possono attivare sul territorio grazie anche e soprattutto all'azione pubblica. Mi riferisco alla delega per il riordino e la semplificazione della programmazione negoziata, che ha esaurito la sua spinta propulsiva degli anni Novanta e che peraltro è stata minore di quella che avrebbe potuto essere se non fosse stata frenata da una normativa un po' farraginosa. Mi riferisco alla semplificazione e al riassetto degli adempimenti procedurali e degli adempimenti richiesti alle imprese e alle misure a favore dell'internazionalizzazione delle imprese e dello *start‑up* di imprese internazionali (internazionali per la localizzazione degli investimenti o per la penetrazione

alla promozione imprenditoriale e all'internazionalizzazione. Mi riferisco alla forte azione a tutela dei marchi e delle denominazioni geografiche e di origine, con giusti inasprimenti delle sanzioni in materia di contraffazioni, sia

misure compensative per le popolazioni ed Agenzia per la sicurezza nucleare, oltre alle misure per le energie rinnovabili. Vorrei spendere un paio di minuti per sottolineare che il provvedimento si occupa anche di trasporti. Lo fa nella logica e nella filosofia che ho cercato di riassumere in questo intervento. Tuttavia, fatte salve le buone intenzioni (che sono al di là di ogni dubbio), in qualche punto tali misure rischiano di produrre un effetto che non è esattamente quello sperato. In particolare, esse vanno un po' controcorrente rispetto al disegno complessivo

riducendola addirittura al solo *incumbent*, l'operatore preesistente), vanificando di fatto la concorrenza. Mi riferisco ad una specifica discriminazione fra operatori italiani e operatori dell'Unione europea, che nasce per rispettare le esigenze di reciprocità di trattamento che in realtà sono tutelate da altra norma e quindi probabilmente non era necessaria. Mi riferisco al fatto che venga indicato il Ministero dei trasporti come soggetto regolatore del mercato, e questo mi pare improprio dal momento in cui in Italia esiste un'istituzione, l'Autorità un'istituzione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che serve esattamente a questo, e soprattutto in considerazione del fatto che il Ministero, proprio nella normativa introdotta, è uno dei soggetti che può chiedere la verifica del danno eventualmente apportato dal nuovo entrante. Quindi, avremmo un Ministero che si fa la domanda e si dà la risposta, che, con tutta evidenza, non è la soluzione

al dettato europeo, così come la possibilità prevista dall'articolo 33-*octies* di procedere ad affidamenti diretti su base regionale, senza precludere all'impresa affidataria la partecipazione a gare in altre Regioni.

di una norma che finalmente stabilisca, fuori di ogni dubbio e coerentemente con la giurisprudenza comunitaria, la necessità di una separazione reale, a livello di imprese, fra gestore dell'infrastruttura e gestore del servizio, e non solo di una separazione formale a livello di società. Questo può essere oggetto

anticipo il mio voto favorevole, anche in caso di eventuale bocciatura degli emendamenti a mia firma, proprio perché il provvedimento costituisce un tassello fondamentale per ricostruire gli standard di competitività e favorire la reale modernizzazione del Paese.

è stato detto da più senatori che siamo di fronte ad un provvedimento stravolto dal lavoro in Commissione.

uso questo termine - fanno ostruzionismo a se stessi in un provvedimento di legge con centinaia di emendamenti presentati e con un lavoro parlamentare nelle Commissioni di merito ostacolato dalla difficoltà della contestuale presenza di numerosi decreti-legge che ne impediscono l'esame in Commissione bilancio. Penso che su questo andrebbe fatta una riflessione. I mesi che ci attendono saranno difficili e mi auguro che non avremo solo da discutere e approvare decreti-legge ma, come in quest'occasione, disegni di legge e quindi provvedimenti di carattere generale che possono dare un contributo. In questo caso parliamo di imprese, di internazionalizzazione, di sviluppo e di energia. Purtroppo il nostro lavoro è stato ostacolato; eppure, non è mancato il contributo che l'opposizione e il Partito Democratico hanno dato anche in questo ramo del Parlamento, così come alla Camera. Ne sono testimoni il

Abbiamo ottenuto importanti risultati in questo lavoro. Quando il Parlamento funziona e viene valorizzato, c'è un risultato positivo da entrambi le parti nel merito delle questioni. Vorrei ricordare alcuni provvedimenti che sono stati migliorati dal nostro punto di vista e che portano il contributo esplicito del Partito Democratico: l'estensione e il rafforzamento dei poteri dell'*Authority* sull'energia e il gas, che credo sia un elemento decisivo nel momento in cui mettiamo mano organicamente alla legislazione nel settore energetico del nostro Paese; il tema del trasporto aereo, in particolare con riguardo ai servizi a terra; il prolungamento del tetto *antitrust* per il gas dal 2010 al 2015 che, mi auguro, la maggioranza non voglia cambiare, come alcuni annunci sembrano voler fare, nel corso del dibattito in Aula. ho trovato un po' stonate le reazioni quasi stizzite del *management* dell'ENI dopo l'approvazione dell'emendamento in materia. Noi siamo non solo per la difesa, ma per la piena valorizzazione dei protagonisti industriali del nostro Paese; non potrebbe essere altrimenti. Quelli che sono i campioni industriali del nostro Paese nell'energia come nell'impresa manifatturiera hanno non solo il pieno sostegno, ma la nostra solidarietà in questa difficile fase della competizione internazionale.

ci sia più efficienza, più sicurezza e più concorrenza, perché di questo si possano avvantaggiare i consumatori e le imprese nel nostro Paese. E poi ancora: l'efficienza energetica; i vincoli abbattuti per il risparmio energetico; gli incentivi alle rinnovabili e così via. Insomma, su tali aspetti abbiamo potuto intervenire e su di essi abbiamo dato un contributo al miglioramento del testo

dal collega Musso un riferimento al trasporto ferroviario. Noi troviamo assolutamente incomprensibile che in un provvedimento che porta per titolo l'internazionalizzazione delle imprese e lo sviluppo dell'energia si inserisca, nel dibattito e nel confronto in Commissione, un maxiemendamento, presentato da un

di una grave scorrettezza istituzionale e di un precedente, caro Presidente, che credo non vada a merito del lavoro del Senato. Parliamo di trasporto ferroviario, di passeggeri, di servizio universale, di trasporto pubblico locale: gli interventi in tali settori avrebbero avuto necessità di essere

dell'energia nucleare. Ho paura - e ho ascoltato interventi in questo senso nel dibattito svoltosi finora - che l'ideologia sia da un'altra parte, ossia nei banchi della maggioranza. Il nucleare è questione troppo seria per essere affrontata in termini ideologici e con forzature non solo nelle procedure, ma anche nel rapporto democratico con le comunità locali e con le istituzioni locali, nonché in materia tecnologica, ed è tale da meritare un approccio diverso da quello che il Governo e la maggioranza hanno inteso riportare nel provvedimento

non ci hanno convinto le motivazioni del ministro Scajola - che, in qualche modo, prefigura quelli che saranno, una volta che tale provvedimento diventerà legge, i requisiti e le tipologie degli impianti che verranno utilizzati in Italia, attraverso un rapporto privilegiato

ad una competizione internazionale che non si è potuta realizzare a causa dell'accordo stipulato tra il Governo italiano e il Governo francese, tra l'ENEL e l'EDF. Di questo stiamo parlando. Avremmo voluto su questo tema e mi auguro che l'Aula possa farlo nelle giornate che verranno. Vorremmo ci fosse un'Agenzia per la sicurezza dotata di poteri reali, di risorse, come è stato detto da altri colleghi del nostro Gruppo; vorremmo che l'Agenzia per la sicurezza avesse a garanzia a garanzia degli italiani, non di una parte di questo nostro Paese, non di una maggioranza o di una parte del Parlamento, quei criteri di terzietà e di autonomia senza i quali nessuno potrà sentirsi garantito di fronte all'industria nucleare. Di questo vorremmo

le fonti rinnovabili sono uno straordinario investimento per il nostro Paese. Provengo da una Regione, la Puglia, che oggi esporta l'88 per cento dell'energia prodotta sul proprio territorio, la gran parte della quale proveniente da fonti rinnovabili, essendo la Puglia diventata ormai da qualche tempo *leader* nel nostro Paese nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò rappresenta un grande investimento capace di produrre ricchezza, occupazione, nuove imprese, innovazione tecnologica, di dare un contributo decisivo alle sorti dello sviluppo del nostro Paese, ma anche al raggiungimento degli obiettivi del cosiddetto protocollo di Kyoto. Vorrei che attorno al tema del risparmio energetico, dell'efficienza, dell'utilizzo intensivo delle fonti rinnovabili non ci fosse un atteggiamento di questo tipo, quasi fossimo di fronte a scelte seconda classe. Siamo di fronte ad una grande rivoluzione industriale e di fronte a noi, in queste settimane, vi è un esempio che sta guidando il mondo

in queste ore, in questi giorni, sta compiendo grandi investimenti, anche in termini di cooperazione industriale (a cominciare dalla Chrysler in America), all'insegna del risparmio energetico e dell'efficienza.

dopo aver seguito in Commissione industria l'esame del disegno di legge n. 1195, mi fa particolarmente piacere intervenire perché ritengo che questo provvedimento, oltre alle tematiche che affronta, abbia il pregio della tempestività in un momento storico di particolare crisi economica. E quale settore, se non l'energia, incide tanto sulla spesa di ogni Paese e di ogni famiglia? Questo provvedimento razionalizza e semplifica una serie di norme in diversi ambiti di intervento e, soprattutto, potenzia il settore energetico attraverso un ricorso alle fonti rinnovabili, all'efficienza ed al risparmio di energia; soluzioni alle quali si deve aggiungere il ricorso al nucleare, su cui mi soffermerò tra un po'. Oggi sappiamo che l'Italia dipende dall'energia importata dall'estero per una percentuale che si aggira intorno all'85 per cento. Ci dobbiamo rendere conto che questo dato è inaccettabile e, pertanto, ben vengano tutte le norme contenute in questo provvedimento che, anche indirettamente, tendono a ridurre tale dipendenza. Riduzione che si può ottenere tramite varie strade: il risparmio, gli incentivi alle imprese, il nucleare e così via. Del 15 per cento dell'energia prodotta dall'Italia, il 70 per cento proviene da impianti a combustibili fossili, il cui impatto ambientale, sommato a quello dovuto ai veicoli da trasporto, agli impianti di riscaldamento e ad altre fonti di inquinamento, causa tutte quelle problematiche ambientali che oggi sotto i riflettori di tutto il mondo. a tal proposito ricordare l'impegno del Parlamento europeo con il pacchetto sul rapporto clima-energia «20-20-20». I *target* di questo pacchetto sono molto ambiziosi, richiedono legislazioni nazionali *ad hoc* e probabilmente degli aggiustamenti a livello europeo. Sarà molto difficile per la Commissione europea raggiungere l'obiettivo senza indicatori intermedi del miglioramento del *target* e senza poterli collegare. Quindi, il presente disegno di legge potrebbe avere il gradito effetto collaterale d'iniziare un circolo virtuoso legislativo ai fini del miglioramento globale della situazione energetica e ambientale, diventando il primo provvedimento di vasto respiro in campo energetico proprio a livello europeo. Ed arrivo al tanto osteggiato nucleare e chiarisco che non parliamo più delle antiquate centrali - lo ha detto anche qualcuno prima di me che, seppur sporadicamente, hanno creato problemi alla popolazione e all'ambiente. Le centrali moderne sono strutture di terza generazione che hanno una ridotta produzione di scorie e consentono notevoli vantaggi nella loro dismissione. Noi ora, nel prevedere la costruzione di centrali nucleari sicure ed ecocompatibili, prevediamo anche norme per la massima sicurezza sia degli addetti ai lavori, che della popolazione che abita le zone che verranno individuate,

e per tutte le norme previste, il disegno di legge è particolarmente benvenuto e ben si inserisce nell'accordo recentemente firmato dal presidente Berlusconi con il presidente Sarkozy. Non voglio dimenticare di dire che, a superamento di ogni necessità futura, viene istituita un'Agenzia per il nucleare che, tra i suoi vari compiti, ha quello di regolamentare e controllare l'utilizzo dell'energia nucleare nonché la gestione dei rifiuti e la vigilanza su tutto il sistema, ambiente compreso. Ritengo pertanto che il peso di questo provvedimento si farà sentire positivamente in più di un campo e avrà ricadute positive sia sulla produzione di energia, sia sulla situazione economica, sia sulla riduzione dell'inquinamento ambientale in Europa. C'è ancora tanto altro da dire perché è stato molto lungo il percorso in Commissione. Anche con il contributo della minoranza abbiamo dibattuto per settimane insieme al Governo.

intervengo per esprimere la mia forte preoccupazione sulle misure contenute nel disegno di legge che riguardano il settore dell'energia. Giustamente l'agenzia di stampa ANSA definisce il tema del nucleare il cuore di questo provvedimento. Questo disegno di legge apre la strada alla costruzione di centrali nucleari con l'argomentazione che l'Italia non possa ulteriormente dipendere dall'importazione dall'estero. Effettivamente, la sfida energetica è molto importante per lo sviluppo economico e sociale non solo del nostro Paese ma di tutto il mondo, che quello industrializzato sia quello in via di sviluppo. energia è destinata a crescere e nello stesso tempo le emissioni di gas aumentano l'effetto serra, con conseguenze drammatiche per il nostro Paese. I prezzi delle materie prime energetiche restano elevati e sono esposti - come abbiamo vissuto negli ultimi mesi - ad un'altissima volatilità risultante da grandi speculazioni. Como sottolinea lo stesso Governo, l'85 per cento del nostro fabbisogno energetico riferito al 2007 viene coperto da energie importate rispetto al 50 per cento della media europea riferita ai 27: Il Governo ora spera di poter risolvere il problema puntando sullo sviluppo dell'energia nucleare e sulla costruzione di centrali nucleari. Il primo passo compiuto è già preoccupante:

«Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di controllo (...) sono svolte da autonomi uffici (...) collocati a livello centrale», e «le amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco». vigili del fuoco». La scelta di secretare le fasi di attuazione del programma nucleare è dettata dalla consapevolezza che la popolazione risponderebbe con la massima ostilità all'insediamento di nuove centrali nei loro territori. Con questa scelta si presenta una svolta radicale a quanto finora perseguito dai Governi italiani dopo il noto *referendum* del 1987. In quella occasione, lo ricordiamo, gli italiani dissero no alla costruzione di centrali nucleari, con un risultato molto netto dell'80,6 per cento dei votanti. Oltre a violare questo verdetto popolare, finora non contrastato da nessuna altra scelta popolare, la domanda che si pone è se il ritorno al nucleare sia una scelta conveniente sia dal punto di vista economico, che da quello tecnico. In verità, questa scelta si presenta come una strada completamente errata, con gravi conseguenze sia per l'attuale generazione, che per le generazioni future. L'energia nucleare non è una soluzione per il futuro: è pericolosa, è costosa, non risolve il nostro problema di dipendenza, è una scelta irresponsabile. Entro nel dettaglio. L'energia nucleare è pericolosa perché anche gli impianti più progrediti non garantiscono la piena sicurezza dal punto di vista tecnico, lasciando sempre un certo margine di rischio (il cosiddetto *Restrisiko*); è dunque pericolosa sia sotto il profilo della radioattività che della proliferazione. Oltre a ciò, le centrali nucleari possono essere facilmente prese come bersagli per eventuali attacchi terroristici e bellici. Oltre ad essere pericolosa, questa scelta è anche costosa. I costi di costruzione delle centrali nucleari sono molto alti. I costi della centrale finlandese di Olkiluoto, per esempio (l'unico reattore di terza generazione evoluta in costruzione nel mondo insieme a Flamanville, in Francia), sono lievitati quasi del 50 per cento: dai 3,2 miliardi di euro previsti ai 4,5 attuali. Oltre ai costi di costruzione ci sono i costi dell'uranio, che stanno crescendo a dismisura. Infatti, nel 2000 un chilogrammo di uranio, costava 7 dollari, mentre oggi ne costa 120. Questa è una spesa che l'Italia, in piena crisi economica, non può davvero permettersi. Il nucleare non risolve poi il problema di dipendenza dall'estero, perché la materia prima deve essere pure importata, dunque passiamo da una dipendenza all'altra. Oltre a Oltre a ciò, la materia prima non è eterna, ma molto limitata. Secondo le stime delle organizzazioni internazionali, l'uranio sarà reperibile solo per pochi decenni. Sappiamo, infatti, che le riserve di uranio, concentrate in Australia e Kazakistan, sono appena sufficienti ad alimentare gli attuali 440 reattori per 40-50 anni. Quindi, le nuove centrali annunciate avrebbero problemi di alimentazione e arriverebbero tardi, come dimostra la vicenda dell'EPR in Finlandia. Il nucleare è inoltre una scelta irresponsabile, perché i futuri rifiuti saranno un peso che devolveremo ai nostri figli. Non devo ricordare in questa sede che in Italia si è presentato come grandissimo problema gestire anche i semplici rifiuti solidi urbani. Oltre a ciò, il nucleare non serve a ridurre i consumi di petrolio, visto che il petrolio oggi è utilizzato soprattutto nei trasporti e negli usi civili, e pochissimo per produrre elettricità.

Tutti campi su cui investono tutti gli altri Paesi europei, *in primis* la Germania, e gli Stati Uniti di Barack Obama. Occorrerebbe favorire misure volte a rilanciare il settore delle energie rinnovabili, come pannelli solari, energia eolica, energia termica terrestre, CasaClima, che in Germania e in Italia, nella Provincia di Bolzano, sono proficuamente in uso. Prima di concludere, mi permetto di evidenziare le misure intraprese dalla Provincia di Bolzano, che ha saputo dimostrare che il nucleare non è la soluzione. Il punto decisivo della nostra politica energetica é il risparmio energetico. Negli appartamenti privati il risparmio può arrivare fino al 90 per cento. Faccio un unico esempio:

Non devo inoltre ricordare il successo che la Provincia ha vissuto con il concetto di CasaClima, conosciuto in tutt'Italia e con cui, per esempio, la nuova Camera di commercio di Bolzano è stata costruita a costo zero, quanto al Per quanto riguarda l'energia alternativa, la Provincia di Bolzano, tra l'altro in una zona climatica molto esposta, in cui il consumo energetico per le caldaie è molto elevato, punta sull'idroelettrico, sulla biomassa, sull'energia solare, sulla pompa di calore e per il futuro conta molto sull'energia geotermica. La nostra Provincia copre attualmente, senza la mobilità, il 54 per cento con energia alternativa

La detraibilità dall'IRPEF degli investimenti per la riqualificazione energetica è ideale (in questo senso faccio i miei complimenti al Governo); noi colleghiamo il progetto casa del Governo Berlusconi alla riqualificazione energetica, cioè solo chi risparmia energia potrà aumentare la cubatura e il sottotetto. Questa politica crea posti di lavoro, è espressione di tutela del clima, aumenta la qualità abitativa, riduce la dipendenza dall'estero, è fonte di sperimentazione. Un Governo responsabile, soprattutto nei confronti delle future generazioni, dovrebbe puntare maggiormente su un futuro sostenibile e promuovere un piano inteso alla salvaguardia di ambiente e biosfera. L'appello che lancio è dunque di puntare finalmente su un'altra politica energetica sostenibile.

si è detto che il provvedimento che ci apprestiamo a votare costituisce un ponte verso il futuro nella materia dell'energia. È vero: noi stiamo discutendo del nostro futuro; stiamo discutendo di quale sarà il il costo della bolletta energetica, estremamente pesante per il nostro Paese; stiamo operando delle scelte ed il dibattito che le accompagna avrebbe sicuramente meritato un'attenzione diversa, perché probabilmente non ci stiamo rendendo conto sino in fondo dell'enorme incidenza di ciò che stiamo per approvare. Fa rabbia pensare che negli Stati Uniti si avvia un programma sull'energia solare termodinamica con il genio italiano, con i progetti italiani. Fa rabbia pensare che Siviglia, nel 2011, sarà la prima città in Europa ad avere energia solare termodinamica al 100 per cento con progetto italiano, con il genio italiano. Fa rabbia pensare che la Libia ha iniziato la costruzione della centrale a ciclo solare termodinamico con un'industria italiana. Fa rabbia pensare che il Governo austriaco, neanche un mese fa, abbia deciso di avviare il progetto per il solare termodinamico; che la Germania abbia stipulato, nel 2008, un accordo con i Paesi nordafricani per le centrali solari termodinamiche. Tutto ciò avviene con il nostro genio e con le nostre industrie. In Italia no. Perché? Perché in Italia non accade? Noi non stiamo parlando di qualcosa di futuristico e di irrealizzato, stiamo parlando di qualcosa che è già realizzato. Gli altri Paesi europei hanno fatto questa scelta e si muovono in questa direzione con decisione. L'Italia no. L'Italia aveva progettato e previsto, con l'accordo Stato-Regioni del 2007, di avviare quattro progetti, in Sardegna, Calabria, Puglia e Lazio, per la costruzione di quattro centrali a ciclo solare termodinamico, progetti abbandonati da questo Governo. Perché?

Ed è un delitto che si sta consumando ai danni del nostro Paese. Questa non è una scelta, è un delitto. Ne risponderemo in futuro quando avremo portato a conclusione questa scelta scellerata, costruendo le centrali nucleari nell'arco di 10-12 anni, centrali che costeranno ognuna non meno di 10 miliardi di euro, quando le centrali solari termodinamiche si costruiscono in due anni e i costi vengono ammortizzati in cinque! Questa è la realtà.

di trattamento delle scorie è il processo di vetrificazione, la cui tenuta viene garantita per 80-100 anni.

si realizzano nel resto del mondo e non in Italia? Perché Carlo Rubbia fu licenziato dal Governo Berlusconi nel 2005, andando a realizzare in Spagna e in Nevada ciò che avrebbe potuto realizzare

altro punto di questo provvedimento, che io ritengo assolutamente offensivo nella logica economica, riguarda le aliquote di prodotto che gli estrattori devono corrispondere allo Stato italiano. Ma per quale motivo

Ciò era comprensibile quando i concessionari erano pubblici, ma ora sono aziende private. Perché tutto il mondo fa pagare il prodotto e noi dobbiamo regalarlo?

dando questo enorme beneficio ai concessionari? Avevamo sfidato il Governo a darci queste risposte

Oggi ci viene proposto questo provvedimento, che io non considero assolutamente nel segno della riscossa del nostro Paese per un futuro economico migliore. Io considero queste scelte, che sono centrali in questo provvedimento (come veniva ricordato), come un delitto che si sta commettendo ai danni del popolo italiano.

ritengo questo provvedimento di straordinaria importanza e sicuramente molto atteso, considerato il particolare momento di crisi economica che stiamo attraversando. Al di là di tutte le iniziative lodevoli che il Governo e il Parlamento stanno attuando a sostegno e rilancio dell'economia, la politica energetica è tra le primarie iniziative che dobbiamo attuare per il rilancio della

tutti, in maniera trasversale, abbiamo ritenuto che l'ambiente sicuramente è uno dei temi principali della discussione politica non solo italiana, ma anche a livello mondiale.

si parla di CasaClima e di impianti fotovoltaici. Anche il senatore Li Gotti ha giustamente fatto un passaggio, anche se meno rilevante, su questo argomento. Condivido pienamente, però, per quanto riguarda il senatore Oskar Peterlini (come sappiamo tutti), egli viene da

quel grandissimo provvedimento che ha appena una settimana e mezza di vita, ossia il federalismo fiscale, finalmente anche tantissimi altri Comuni potranno tenersi le risorse nel proprio territorio e investire in energia pulita, in energia alternativa. In

molto lungimirante perché porterà un notevole beneficio a tutti i Comuni medio-piccoli. Sappiamo, da ragionamenti e da ricerche che abbiamo condotto, che, per quanto riguarda i bilanci dei Comuni medio-piccoli, la spesa dell'energia elettrica si aggira su una percentuale che va dal 5 al 7 per cento. Riuscire a produrre in proprio l'energia elettrica significa risparmiare

le casse comunali che in questo momento - come sappiamo - sono abbastanza vuote, in attesa chiaramente di quel federalismo fiscale che abbiamo approvato

finestra"). Onorevoli colleghi, come precedentemente convenuto, anche in linea con quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, ricordo che domani mattina, conclusa la discussione generale sul disegno di legge collegato, si svolgeranno le repliche del relatore e del Governo. Si passerà quindi alla discussione del disegno di legge sull'ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità. Durante la trattazione di tali argomenti da parte dell'Assemblea, la 5a Commissione potrà proseguire, in sede consultiva, i propri lavori

recentemente, ho aderito all'invito di parlare al termine, anche se devo dire che diventa un po' diverso. Signor Presidente, domenica scorsa in Afghanistan si è verificato un tragico evento: una ragazzina di 13 anni afghana è stata uccisa ad Herat. Il Comando italiano nella regione ha segnalato che i nostri militari hanno fatto fuoco dopo aver attuato tutte le procedure di segnalazione previste. Sappiamo che sono in corso due inchieste, dei Carabinieri italiani e della Polizia afghana, per appurare lo svolgersi dei fatti e per capire come si sia potuto verificare questo tragico incidente. Resta il dramma di una giovane vita spezzata e di alcuni feriti tra i familiari. Resta, d'altro canto, il ruolo importante che i nostri militari stanno svolgendo in quei territori in cui, fino ad oggi, sono stati riconosciuti per aiutare la popolazione secondo il senso della nostra missione internazionale.

Fino adesso l'atteggiamento della popolazione è sempre risultato di positivo apprezzamento per il grande lavoro e l'impegno profuso dai nostri militari e quindi per il nostro Paese. Credo dunque doveroso che, oltre ad esprimere i sentimenti di cordoglio dell'Aula del Senato alla famiglia della bambina (al riguardo, mi permetta, Presidente:

Grazie